nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio si è svolto un ciclo di audizioni che ha consentito di acquisire elementi istruttori sul punto di vista delle parti sociali e dei soggetti istituzionali. Sono stati acquisiti i pareri di tutte le altre Commissioni permanenti; il Governo ha fornito chiarimenti sulle richieste informative del Parlamento; i Gruppi hanno espresso le rispettive posizioni e, infine, la Commissione mi ha conferito il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea (DEF) 2023, sulla Relazione annessa e sugli altri allegati. Il Documento di economia e finanza rappresenta il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica del Paese, previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica. La prima sezione del DEF reca lo schema di programma di stabilità; la seconda sezione riporta l'analisi e le previsioni dei dati di finanza pubblica a legislazione vigente; la terza sezione, infine, la terza sezione, infine, espone il programma nazionale di riforma. Dopo l'esame parlamentare, il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma verranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, il DEF espone il quadro relativo all'anno 2022 e le previsioni tendenziali e programmatiche per gli anni fino al 2026. Le previsioni del quadro macroeconomico tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica di bilancio messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF stesso. Il quadro programmatico include invece l'impatto sull'economia delle politiche economiche che saranno concretamente definite nella NADEF di settembre 2023 e adottate con la prossima legge di bilancio. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in data 7 aprile 2023, mentre il quadro programmatico è stato validato nell'audizione del successivo 20 aprile. Richiamando le stime ufficiali dell'Istat, il Documento evidenzia come il PIL abbia registrato nel 2022 una crescita del 3,7 per cento in termini reali, in linea con quanto prospettato nel Documento programmatico di bilancio del novembre scorso. Sulla base dell'andamento congiunturale, in considerazione del miglioramento del contesto internazionale dovuto a un calo dei prezzi energetici più rapido delle attese, le prospettive per l'anno in corso risultano moderatamente più favorevoli rispetto alle previsioni ufficiali contenute lo scorso novembre nella NADEF. Nello scenario tendenziale a legislazione vigente il PIL per il 2023 è pertanto previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento, in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico della NADEF. Per quanto riguarda gli anni successivi, la previsione di crescita del PIL per il 2024 è prevista all'1,4 per cento, più sostenuta rispetto al 2023, ma al ribasso rispetto all'1,9 per cento previsto nella NADEF, essenzialmente a causa del peggioramento delle variabili esogene. La crescita per il 2025 resta invece invariata all'1,3 per cento, come già previsto nella NADEF. La previsione per il 2026 viene posta all'1,1 per cento, convergente verso il tasso di crescita potenziale dell'economia italiana stimato secondo la metodologia definita a livello europeo.

Venendo alla sezione del DEF dedicata agli andamenti di finanza pubblica, i dati riferiti all'anno 2022 attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a 151,9 miliardi di euro, corrispondente all'8 per cento del PIL, superiore al livello del 5,1 per cento previsto nella NADEF. Per quanto attiene al quadro previsionale a legislazione vigente, il conto economico evidenzia per il 2023 un indebitamento netto pari al 4,4 per cento del PIL. Per gli anni successivi si stima un costante decremento dell'indebitamento netto sia in valore assoluto, sia in rapporto al PIL, nei seguenti termini: 84,8 miliardi nel 2024, 70,5 miliardi nel 2025, 67,8 miliardi nel 2026. L'indicata evoluzione dell'indebitamento netto è determinata principalmente dal miglioramento del saldo primario, il quale in rapporto al PIL migliora in tutti gli anni del quadriennio, passando dal -0,6 per cento del 2023 al +2 per cento del 2026. A ciò si accompagna tuttavia un aumento della spesa per interessi, che, sempre in rapporto al PIL, passa dal 3,7 per cento nel 2023 al 4,5 per cento nel 2026. Per quanto riguarda il quadro programmatico di finanza pubblica, il Governo evidenzia che la politica economica impostata è coerente con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea con riferimento alla necessità di continuare ad attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi energetici sulle famiglie e sulle imprese, mirando al contempo a ritirare gradualmente le misure adottate man mano che i prezzi si stabilizzano, coerentemente con una gestione prudente della finanza pubblica. del Governo è quello di sostenere la domanda privata e contrastare il calo del potere d'acquisto delle retribuzioni causato dall'inflazione. Alla luce di quest'orientamento e del miglioramento della previsione d'indebitamento netto tendenziale,

Per quanto riguarda l'evoluzione del rapporto debito pubblico-PIL, la stima preliminare per il 2022 indica un livello del 144 per cento, inferiore al livello del 145,7 per cento previsto dalla NADEF 2022 2022 del novembre scorso. Il risultato migliore rispetto alle stime viene spiegato dal DEF con la maggiore crescita economica e con un andamento dei saldi di cassa migliore delle attese. Il fabbisogno del settore pubblico a fine 2022 si è attestato infatti al 3,4 per cento del PIL, anziché al 4 per cento atteso a novembre. Quanto alle previsioni, il DEF stima il rapporto debito-PIL in riduzione anche nell'anno corrente e nei tre successivi. Infatti, pur in un quadro d'incertezza legato alla guerra in Ucraina e alle pressioni inflazionistiche, la componente legata alla crescita del tasso d'interesse dovrebbe contribuire alla riduzione del rapporto debito-PIL per effetto di una sostenuta crescita economica e di un'elevata inflazione, che compenserebbero l'aumento dei tassi di interesse. In particolare, nel 2023 nel 2023 il DEF prevede un rapporto debito-PIL pari al 142 per cento, in riduzione rispetto al 2022. A completamento della manovra di bilancio, nel DEF il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio ventuno disegni di legge, i primi tre dei quali già presentati presso uno dei due rami del Parlamento. Al DEF 2023 sono inoltre allegati sei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si rileva inoltre che la relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile per il 2023 è stata pubblicata in data 2 marzo 2023 e successivamente trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Si segnala infine che l'articolo 22-*bis*, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che sia allegata al Documento di economia e finanza una relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri, la quale non risulta al momento presentata. Unitamente al DEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine, ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'obiettivo di medio termine (OMT) siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Con la Relazione presentata come documento annesso al DEF 2023, il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici, più favorevole negli anni 2023 e 2024 rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissato per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022. In base a quanto riportato nella relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento, pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024, saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzata a sostenere il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, limitando al contempo la rincorsa salari-prezzi, in particolare attraverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.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 Signor Presidente, nella premessa al DEF il ministro Giorgetti sottolinea come il Documento sia prudente e mostri una "immutata coerenza" queste sono le sue parole - per aver confermato gli obiettivi di *deficit* pubblico fissati sei mesi fa. Permettetemi di dissentire da quest'affermazione. Partiamo dalla questione della coerenza rispetto agli obiettivi annunciati sei mesi fa: essa è soltanto apparente, perché gli obiettivi di *deficit* per il 2023 e per gli anni seguenti sono immutati,

di riclassificarli. Per essere davvero coerenti in termini di accumulo di debito pubblico, in particolare, sarebbe stato necessario rivedere verso il basso gli obiettivi di *deficit* per il 2023 e gli anni seguenti (questo, in termini di coerenza). non contiene l'indicazione di quanto, anno per anno, i *deficit* per il 2023 e gli anni seguenti siano stati sgravati, il che sarebbe stato invece molto utile, ma informazioni ricevute informalmente indicano che si tratta di 4 miliardi quest'anno e di ben 16 miliardi nel 2024. Ciò significa che - attenzione - utilizzando lo stesso criterio di contabilizzazione dei *bonus* edilizi usato sei mesi fa,

del 4,5 anziché del 3,7. Insomma, è una coerenza totalmente fittizia. In realtà, si stanno indebolendo gli obiettivi di *deficit* pubblico. Uno potrà essere d'accordo o meno sul farlo o no, ma per queste cifre indebolendo gli obiettivi di *deficit* pubblico. La diversa classificazione dei *bonus* edilizi ha un'altra conseguenza. Lo spazio di manovra tra *deficit* programmatico e tendenziale, incluso nel DEF e utilizzato per questo tesoretto della piccola manovra espansiva, è del tutto fittizio: al netto dello spostamento contabile dei *bonus* edilizi, il tendenziale per il 2023 sarebbe uguale al programmatico nel 2024 il tendenziale sarebbe più alto del programmatico dello 0,6 per cento del PIL, il che richiederebbe - per essere coerenti - una manovra correttiva nel 2024 di ben 12 miliardi, il piccolo tesoretto che il Governo dice di ritrovarsi è dovuto puramente a una riclassificazione contabile. La riclassificazione dei *bonus* nasconde un altro fatto preoccupante su cui il DEF non si sofferma: al netto della riclassificazione, il *deficit* tendenziale primario quest'anno è di 8 miliardi peggiore di quanto programmato sei mesi fa, un indebolimento che sale a 10 miliardi nel 2024. Il DEF non spiega a cosa è dovuto questo indebolimento: lo abbiamo chiesto in audizione al Ministro, ma non è arrivata risposta. Non abbiamo avuto risposta chiara in audizione neanche su un altro aspetto. Nel 2023 la spesa per interessi è misteriosamente prevista in calo di 8 miliardi circa rispetto alle previsioni fatte soltanto sei mesi fa,

Il Ministro in Commissione ha detto che questo è dovuto alla minore inflazione rispetto a quanto previsto, il che influisce sulla spesa dei titoli indicizzati per un importo corrente, ma il DEF ha un'inflazione più alta di quanto era stato previsto sei mesi fa, quindi il mistero resta. Questa è un'altra cosa che non si capisce. Passo all'andamento del debito pubblico. Il Governo ritiene, ovviamente, che il quadro di riduzione del debito sia adeguato. Tuttavia, la riduzione del debito pubblico nel quadro è dovuta solo alla tassa d'inflazione che grava sui risparmiatori:

il rapporto tra debito pubblico e PIL quest'anno, anziché scendere, aumenterebbe di almeno un punto percentuale di PIL, anche ipotizzando tassi d'interesse più bassi. Anche nel 2024 ci sarebbe un piccolo aumento, che diventerebbe più sostanzioso - oltre un altro punto percentuale - se la crescita, anziché accelerare, come previsto cosa di per sé molto incerta - continuasse al ritmo previsto per quest'anno. Quindi, anche i dati del debito vanno bene, ma soltanto perché si stanno tassando, con una tassa occulta, i risparmiatori. Al di là del 2024, con l'inflazione ritornata al 2 per cento, il processo di riduzione del debito si interrompe quasi completamente, cosa preoccupante anche alla luce della prossima riattivazione delle regole europee sui conti pubblici. In questo contesto, diventa irrealistico permettere sostanziali riduzioni del carico fiscale, posticipi dell'età di pensionamento, aumenti della spesa per Difesa e natalità come nei piani del Governo, tanto meno i piani del Governo possono essere coerenti con quegli aumenti di risorse per sanità e pubblica istruzione che invece sarebbero prioritari. Gli spazi di bilancio sono strettissimi - anzi inesistenti - quando invece potrebbero essere ampliati attraverso una seria lotta all'evasione fiscale e un'attenta revisione della spesa evitando i tagli lineari che sono stati ottenuti negli ultimi due anni, anche in questo caso attraverso l'inflazione. Riguardo all'evasione fiscale, abbiamo avuto i condoni della legge di bilancio e ora una legge delega sul fisco tutta preoccupata di non disturbare troppo gli evasori.

Tutto sommato, con tutto il rispetto e la solidarietà che ho per il difficile lavoro che il Ministero svolge, credo veramente che si potesse fare meglio in termini di coerenza, prudenza e anche trasparenza del DEF.

senatore Calandrini, che ringrazio per il lavoro che ha fatto insieme a tutta la Commissione, ci ha descritto i contenuti del Documento di economia e finanza e gli obiettivi che questo Documento si prefigge, in un in un quadro che chiaramente sottolinea non solo quello che materialmente è scritto, ma che prevede anche una visione e un contesto che si inseriscano in uno scenario internazionale molto particolare: viviamo ancora l'instabilità molto evidente dovuta alle conseguenze della pandemia

Il PIL nel 2022 è aumentato del 3,7 per cento, come ci veniva ricordato; cresce nel 2023, crescerà nel 2024, crescerà nel 2025, crescerà nel 2026. Al contrario, il debito della pubblica amministrazione scende e scenderà quest'anno, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, accanto a quello che il Governo si sta prefiggendo di fare, con una riduzione fiscale e un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti, tutte misure che poi prenderanno vigore nel Consiglio dei ministri che già è stato annunciato per il 1° maggio. Dico questo perché vorrei sottolineare come in questi mesi di Governo del centrodestra lo *spread* sia sceso di centinaia di punti, perché la borsa ha avuto un aumento di circa il 20 per cento, dato che la Banca d'Italia - e non il centro studi di Fratelli d'Italia - ha stimato che l'Italia sarà in netta ripresa quest'anno e la ripresa si stabilizzerà nel 2024 e nel 2025.

prefigurava nel caso di vittoria del centrodestra alle elezioni. Evito per carità di Patria di ricordare i nomi, ma ricordo che qualcuno aveva detto: se vince, la destra ci manda in bancarotta; se vincessero Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, si arresterebbe ogni possibilità di progresso. Queste, rispetto alle cifre che abbiamo appena raccontato e a quello che il DEF ci illustra, erano le previsioni che qualcuno voleva raccontare agli italiani.

signore, ex Ministro, diceva che con il Governo di centrodestra avremmo sfasciato i conti, messo a rischio i risparmi degli italiani, isolato l'Italia in Europa e fatto saltare i fondi del PNRR. Rischiavamo, cioè, secondo lui, «una guerra economica, una catastrofe dagli effetti devastanti», parole testuali.

il «Washington Post» ci dice che la Meloni ha sfidato i profeti di sventura, soprattutto quelli al di là dei confini italiani, e sorpreso i critici e che il suo successo potrebbe diventare un modello per altri politici in Europa. Il Presidente del Consiglio europeo, di cui tanto avevamo paura nei confronti dell'Unione europea, ci dice che c'è stata fino ad ora una cooperazione basata sugli interessi italiani, ma anche sulla volontà di tutelare l'Unione europea: quando sta bene l'Italia, sta bene anche l'Unione europea. Una fondazione di Washington, Heritage foundation, dice che quello presieduto da Giorgia Meloni è uno dei Governi italiani più stabili e attivi da qualche tempo a questa parte, con implicazioni per gli affari europei e transatlantici.

una serie di misure, prevede le risorse annunciate, il risanamento del debito, l'aumento del PIL, ma ciò che è più importante è che rappresenta - come sempre per chi fa politica - una visione. Su questa visione ci sono state tante polemiche, ricordiamo le scelte che sono state fatte. Ricordo la polemica su quando non siamo intervenuti sul prezzo della benzina per aiutare famiglie e imprese; poi, il prezzo della benzina è sceso e le famiglie e le imprese forse stanno meglio; o immagino quando è stata presa la decisione a livello europeo di imporre un tetto unico al gas, motivo per cui oggi il prezzo del gas scende. Vedo anche che si discute finalmente del Patto di stabilità in Europa, dove c'è finalmente più flessibilità, anche grazie a una misura e, se volete, anche a una concezione politica e culturale che portiamo avanti, contrariamente ai Paesi rigoristi. In conclusione, Presidente, a chi vede sempre tutto nero, ai campioni del pessimismo, a chi ci ricorda che il bicchiere è sempre mezzo vuoto e a chi fa il professionista della sventura, ricordo semplicemente che questo Governo, anche grazie al DEF, ha adottato provvedimenti con entusiasmo e con orgoglio, potendo e volendo riportare l'Italia lì dove si merita: ritornare a essere un Paese efficiente e capace, che sappia essere protagonista in Europa e nel mondo.

colleghe e colleghi, signora Sottosegretaria, mi dispiace che il ministro Giorgetti non sia potuto intervenire oggi, non solo per l'importanza assolutamente centrale del Documento di economia e finanza, ma anche perché questi sono giorni di vero crocevia, di decisioni importanti ed estremamente interessanti che si prendono sul piano europeo e sul piano italiano. Sarebbe stato quindi molto interessante avere la visione complessiva del Ministro in questa particolare circostanza. La mia valutazione sul DEF è tendenzialmente positiva: mi sembra ispirato a principi di responsabilità finanziaria. Certo, mi auguro che la Sottosegretaria vorrà rispondere alle considerazioni, come sempre molto pertinenti, del senatore Cottarelli - di cui parlo

venivano diffuse infauste e letali previsioni per il destino della finanza pubblica italiana, ove mai la coalizione guidata da Giorgia Meloni avesse vinto le elezioni. Io non mi sono mai associato in quell'epoca a questa visione. Spesso interpellato da osservatori italiani o stranieri, ho sempre detto che ci se i partiti componenti quella coalizione si fossero attenuti ai principi che hanno spesso esposto, e anche praticato, di scarsa responsabilità finanziaria, ma ero convinto che, una volta al Governo, una volta doppiato il momento delle elezioni, avrebbero spiegato ai cittadini che era iniziato un altro momento e che occorreva un diverso atteggiamento verso la realtà e la serietà, ivi incluso in campo finanziario. Sono stato anche il primo a rilevare che, poco dopo l'ingresso dell'attuale Governo, lo *spread* era sceso di una trentina di punti rispetto a com'era alla fine del Governo precedente.

con soddisfazione l'arrivo di tutti - direi proprio di tutte le parti politiche, a questo punto - a una visione non rigoristica, non macabra, ma seria e solida della responsabilità finanziaria. Forse un partito che nel 2018 ha condiviso il Governo con un altro partito non ha ancora fatto questo passo,

ha invertito una rotta tenuta da alti esponenti del suo partito ancora a Governo Meloni già iniziato e ha dato enunciati con pragmatismo lombardo, rivendicando - ha fatto piacere anche a me

conclusioni che anch'io mi sento di condividere; ha invitato infatti a non dimenticare che, nel caso dell'Italia, due terzi delle risorse che l'Europa è pronta a darci sono prestiti, non *grant*, non sovvenzioni che non sappiamo ancora bene quale sarà il tasso d'interesse da pagare, che ci saranno le rate di rimborso del capitale, il tasso di interesse e di fronte a un'opera che riceve un finanziamento, che però poi non rispetta le scadenze volute dal piano, l'Italia dovrà rimborsare il finanziamento e poi terminare le opere a proprie spese. parole intrise di responsabilità finanziaria, che avrebbe potuto pronunciare qualcuno che anni fa sarebbe stato tacciato di becera e bieca filoausterità. Ben arrivati tutti a questa nuova piattaforma che, parlando del crocevia con le decisioni europee, è molto benvenuta, soprattutto perché entrerà presto in vigore - non sappiamo esattamente quando e soprattutto in quale forma - la nuova formulazione del Patto di stabilità e di crescita,

fare brutta figura domani, perché non è riuscita a fare realmente e produttivamente quel coacervo di cose che a piene mani, e con un certo atteggiamento del pulcino a bocca spalancata che aspetta l'arrivo del genitore, ha chiesto all'Europa - dovesse fare una valutazione pacata, che mi pare sia in corso, che dovesse portare alla conclusione che alcune opere non sono da eliminare o cancellare, ma per tempi, modalità e possibilità alternative di finanziamento è meglio che non facciano parte di questa lista, un po' precipitosamente compilata in passato, io questo lo sottoscriverei. Spero che non ci siano contrapposizioni e polemiche sterili, che non devono più far parte di questa nuova stagione: benvenuti tutti finalmente a questa nuova stagione di responsabilità finanziaria, tra chi dice

Spesso sono stato critico; certamente, ho ricevuto molte più critiche di quante ne abbia emesse nei confronti del sistema politico e parlamentare di questi ultimi dieci-quindici Spesso sono stato a mia volta critico. Vi prego di non perdere di vista che, al di là delle differenti sfaccettature e diverse ricostruzioni del passato, questo, tra ieri e oggi, è un momento non dico storico (si abusa spesso di questo aggettivo), ma significativo, in cui - non so quanto rendendosene perfettamente conto attori importanti hanno scritto una nuova pagina della convivenza italiana in materia finanziaria, che sembra arida e tecnica, ma si chiama semplicemente rispetto dei nostri figli e dei nostri nipoti. Un'ultima considerazione, Presidente: forse c'è ancora una tessera di questo mosaico, che si sta componendo con inaspettato equilibrio e armonia. È quella del MES, che in passato è stato oggetto dei giocolieri più spregiudicati, che ne hanno falsificato le origini storiche e cantato le virtù malefiche. Sembrava Sembrava uno strumento finanziario vicino al mondo delle streghe, da bruciare. Bene, io credo che sia l'ultimo passo che ci resta da compiere verso la razionalità.

la Lega lo accolse con cartelli pittoreschi e molto critici.

e demitizzata considerazione del MES - per evitare che in Europa si pensi che l'Italia sta facendo inaspettati passi verso la responsabilità, ma le rimane un doppio, terzo o quarto pensiero da usare, chissà quando, verso i *partner* europei - è un passo che solleciterei, rallegrandomi

odierna ci apprestiamo ad approvare il primo Documento di economia e finanza di questo Governo di centrodestra. Come sottolineato da tanti colleghi delle opposizioni, forse è anche il primo Governo politico Già da qui nasce la prima riflessione, perché ciò pare sottolineare che chi ha governato negli ultimi dieci o quindici anni è stato in qualche modo orientato nell'agire dalle istituzioni di livello superiore. Detto tra noi, appare più una giustificazione che una realtà. Forse sarebbe più corretto dire che, finalmente, governa chi è stato scelto dai cittadini italiani.

per mettere in sicurezza il Paese e ai fattori che incidono sulla scelta delle azioni da mettere in campo. Come ricordava il senatore Monti, certamente c'è bisogno di responsabilità e bisogna amministrare tenendo presenti anche le risorse che abbiamo a disposizione, stando attenti ad avere un margine, perché gli eventi che si sono succeduti negli ultimi anni non erano prevedibili, ma forse si potevano affrontare in maniera migliore

in Ucraina e l'elevato livello di inflazione che ne è seguita, nonché i recenti episodi di dissesto bancario negli Stati Uniti e in Svizzera, che hanno inevitabilmente alimentato la volatilità sui mercati finanziari, e la crisi idrica.

Questi sono aspetti che non possono farci esultare, perché vogliono dire che il nostro Paese era altamente deficitario. È evidente che chi ha governato negli anni precedenti non ha avuto una visione attenta infatti, negli ultimi anni, si è dovuto ricorrere a una politica di sostegni e *bonus*, per ovviare a queste carenze di visione. Fortunatamente l'Italia è un Paese resiliente, fatto da imprese grandi e piccole che hanno saputo affrontare questo momento e da quel patrimonio di risparmi a cui gli italiani hanno hanno attinto e stanno attingendo e che permettono di sostenere l'economia in questo momento. Difatti, anche l'andamento del PIL e il fatto che non siamo andati in recessione sono dovuti proprio a questo patrimonio, dovuto alle incertezze date dai Governi precedenti, che ponevano gli italiani in condizione di trattenere le risorse in banca piuttosto che spenderle; questa incertezza ha garantito in questo momento risorse indispensabili da rimettere nell'economia reale, che sono state importanti per la ripresa economica del Paese. Questi segnali incoraggianti provengono dalla fiducia delle imprese e delle famiglie e dall'aumento degli indici dei direttori degli acquisti, tornati in tutti i settori sopra la soglia, che corrisponde appunto a un'espansione dell'attività. Bisogna tener conto del Patto di stabilità, che è stato sospeso nel marzo 2020 per lo *shock* economico del Covid, ma che sarà ripristinato nel gennaio 2024. 2024. Risulta necessario rivedere il quadro delle regole europee in materia di *governance*, che si sta discutendo adesso in Europa, perché sarebbe irrealistico tornare a quelle precedenti. Sebbene risulti all'attenzione di tutti il tema della necessaria della necessaria sostenibilità del debito pubblico degli Stati membri dell'Unione europea e della promozione della crescita attraverso investimenti e riforme strutturali, emerge comunque la necessità di una maggiore attenzione alla programmazione programmazione di medio termine, anche nella sorveglianza di bilancio, che tenga conto delle esigenze di ciascuno Stato membro nell'ambito della propria programmazione di bilancio. Nella comunicazione del 9 novembre 2022 si prevedeva che i singoli Stati membri potessero adottare percorsi di aggiustamento della finanza pubblica più graduali, a fronte di precisi impegni per le riforme o investimenti (sette anni Un così ridotto tempo di aggiustamento rispetto all'assunzione di impegni di riforma e investimenti potrebbe essere gravoso dal punto di vista della finanza pubblica, sempre poco adatto ad incentivare i singoli Stati membri. Potrebbe verificarsi che soltanto i Paesi con elevati margini finanziari riescano riescano ad avviare le riforme e gli investimenti necessari. Siamo preoccupati per la proposta della Commissione europea sul nuovo Patto di stabilità, perché avevamo chiesto con forza l'esclusione delle spese di investimento del PNRR dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri. È evidente che, quando si investono

Però ci sono alcune criticità che, quando siamo andati al Governo, ci siamo trovati ad affrontare. Ieri sentivo in Commissione le critiche di alcuni colleghi ai tagli sulla sanità. Ricordo che

Le facoltà di medicina a numero chiuso hanno portato tanti dei nostri studenti ad andare a formarsi all'estero e questo lo paghiamo adesso. Quando parliamo di fuga dei cervelli, dobbiamo anche pensare a come abbiamo agito negli anni passati. Io sono qui dalla scorsa legislatura e mi ricordo che le borse di studio per gli specializzandi erano ferme a quota 8.000. In questi anni sono state incrementate,

risorse devono essere ripristinate in parte dalle Regioni e in parte dalle aziende, mettendo così in crisi un settore strategico e importante per la salute dei cittadini come quello dei dispositivi medici. Un altro tema che stiamo affrontando è quello della crisi idrica. Com'è stata affrontata negli anni passati? Adesso lo stiamo facendo in maniera strutturale, ma ricordo che in una passata legge di bilancio

secondo i dati Istat, infatti, su un totale di 8,2 miliardi di metri cubi di acqua immessa nel sistema, la perdita si aggira intorno ai 3,4 milioni, un dato che corrisponde ad altri 150 litri di acqua sprecata ogni giorno per abitante. Come ha risposto il Governo giallorosso? Con un *bonus* rubinetti di 1.000 euro per sistemare i rubinetti. E poi venite a dire a noi che bisogna essere programmatici e strutturali, e che non abbiamo la responsabilità di governare questo Paese? Credo invece che gli italiani

apre una nuova finestra"). Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Fucini-Roncalli» di Gragnano, in provincia di Napoli. Signor Presidente, membri del Governo, il Documento di economia e finanza (DEF) è il principale strumento di programmazione economica e finanziaria del Paese e definisce gli obiettivi da raggiungere tramite le riforme. Fornisce, in pratica, tutti gli elementi che concorrono alla strategia con cui questo Governo vuole modellare il futuro economico dell'Italia e degli italiani. Ebbene, signor Presidente, dopo aver analizzato bene il DEF del 2023, il grande assente è proprio il futuro. Sì, perché i numeri della crescita del PIL da prefisso telefonico sono avallati dall'immobilismo e da quella politica dei tagli che questo Governo ha operato. Sono tagli che certamente piaceranno ai falchi del Nord Europa, ma molto meno agli italiani, ancora alle prese con un'inflazione del 7,7 nel mese di marzo, che abbassa notevolmente il potere d'acquisto. Questo dopo due anni di crescita del PIL a doppia cifra, grazie agli investimenti e a politiche di sostegno al reddito messe in campo dai Governi Conte I e II. signor Presidente, non viene garantito dall'erosione del numero delle imprese giovanili, su cui questo Documento non fornisce alcun riferimento e che denota, così come nella legge di bilancio, una mancata politica industriale. industriale. Da soli, questi elementi forniscono il quadro di un'Italia in affanno, con gli italiani impegnati a sbarcare il lunario con le rate dei mutui alle stelle e la mancanza di interventi economici e sociali di sostegno al reddito e all'occupazione: uno scenario che scoraggia qualsiasi proiezione del futuro. Eppure, nelle ultime settimane uno dei temi su cui tanto ha discusso questo Governo è stato la denatalità. Ebbene, ricorrendo alla saggezza popolare, viene da dire che non c'è bisogno della zingara per indovinare che uno dei motori principali per invogliare una coppia ad avere figli è avere una prospettiva di futuro e di crescita. Non aiuta la scelta del Governo di aver eliminato il reddito di cittadinanza e, quasi dopo sette mesi, di non aver presentato una misura alternativa di sostegno al reddito. Non aiuta aver tagliato le pensioni in legge di bilancio: ora nemmeno più i genitori e i nonni possono aiutare questi giovani. Non aiuta aver tagliato i fondi per la sanità pubblica e nemmeno la prospettiva di non avere asili nido nei Comuni per l'incertezza dei fondi del PNRR. Mi permetta, Presidente: non basteranno i 15 euro in più in busta paga, per chi una busta paga la percepisce ancora, previsti con il taglio del cuneo fiscale per soli sette mesi. E converrà con me, Presidente, se resto sgomento quando leggo dalle colonne dei giornali che la probabile soluzione contro la denatalità per questo Governo di destracentro sia vietare la fornitura gratuita della pillola anticoncezionale.

è sostanzialmente una fotografia, un accontentarsi dell'andamento e dello scorrere delle previsioni che più o meno erano determinate già negli anni scorsi, con l'avvento del PNRR e con le soluzioni che c'erano;

ma il calo dell'inflazione - come noto - non riporterà i prezzi alla situazione precrisi. Lo vediamo già nel settore edile e in quello delle aziende energivore, che continuano a dare l'allarme e a segnalare la difficoltà di mantenere gli impegni presi e la risposta produttiva necessaria. Soprattutto, se guardiamo seriamente i dati sull'inflazione e la differenza tra ciò che è inflazione riferita al costo del prezzo dell'energia e ciò che invece è inflazione ormai consolidata sui prezzi dei beni di consumo, *in primis* dell'alimentare, ci rendiamo conto che dobbiamo parlare seriamente delle questioni sociali e del potere d'acquisto delle famiglie, perché in realtà stiamo parlando, dopo la fiammata inflazionistica dell'anno scorso e l'assestamento che continua ad esserci quest'anno, di povertà del lavoro e di povertà dei salari.

Nel contempo, come ben sapete, i salari sono aumentati al massimo di due punti. Certo, ci sono stati gli aiuti, quelli dei vari decreti che si sono succeduti in questo periodo, ma conosciamo anche la loro breve durata e, in qualche caso, i ritardi nelle erogazioni. forse non bisogna solo guardare i numeri del PIL e della sua relativa crescita, perché in realtà dietro di essi continuano la divaricazione sociale e una differenza tra chi se la cava e migliora le sue condizioni e le persone che lavorano o che cercano lavoro,

si avvereranno, purtroppo, le preoccupazioni che derivano dall'intervento sul PNRR, cioè l'abbandono delle Case di comunità e delle scelte d'investimento sulla sanità territoriale; in secondo luogo, ci vorrebbero risorse.

per cento del 2023 ovviamente non copre l'inflazione, nel 2024 pensate di ridurlo, il lieve aumento del 2025 e del 2026 continua a dirci - anzi lo dite voi stessi - che ci porterà nel 2026 ad avere una spesa del 6,2 molto meno del rapporto tra spesa sanitaria e PIL che servirebbe per garantire quel livello di Servizio sanitario nazionale che dovremmo garantire al Paese. Potremmo poi parlare di previdenza, ma non saprei bene cosa dire, perché c'è il nulla; c'è la smentita delle tante promesse che avete fatto in fase elettorale non vorrei ricordarvi cos'avete detto sull'adeguamento delle pensioni, in particolare di quelle più basse. Nonostante tutte queste premesse, in realtà c'è una domanda: quando avverranno queste cose? Nelle previsioni di questo triennio non ci sono,

in famiglie monoparentali e che hanno il problema di conciliare la possibilità di lavorare con l'allevamento dei figli, ma intanto neghiamo loro gli asili nido e quindi garantiamo che non possano superare questa difficoltà.

finte aperture che sono state fornite nella discussione sulla legge di bilancio, vorrei ricordare i lavoratori fragili, che continuano tuttora a faticare per riuscire a mantenere il loro posto di lavoro e nello stesso tempo garantirsi la condizione di salute, anche per aspetti i cui costi sono davvero molto relativi. Penso allo *smart working*, che richiederebbe semplicemente la voglia di andare incontro alle persone e di porsi i problemi sociali, non certo di cambiare i bilanci.

Nei provvedimenti collegati al Documento di economia e finanza ci avete annunciato che il 1° maggio, invece di farci festeggiare il lavoro, farete un decreto sull'ulteriore precarietà del lavoro stesso. *(Applausi)*. Credo che non sia questa la strada per poter affrontare né il tema del lavoro, né quello della denatalità. Proprio per questo credo che dobbiate avere invece il coraggio di affrontare la questione salariale, partendo dal tema dell'assenza nel DEF delle risorse per il rinnovo dei contratti collettivi dei lavoratori pubblici, pubblici, dalla necessità delle assunzioni, dal fatto che se continuate a raccontare che le imprese si possono lasciar fare i lavoratori diventeranno sempre più poveri poi potrete anche raccontare loro un minimo di cuneo fiscale, ma soprattutto dovreste spiegare loro perché continuano a essere i maggiori contribuenti dello Stato italiano, mentre per chi ha molto si continua a dire che bisogna ridurre la pressione fiscale.

una parola più di ogni altra identifica e qualifica il Documento di economia e finanza che il Governo ha presentato alle Camere: svolta. È un documento di svolta, una svolta coraggiosa, ambiziosa, ma estremamente lucida e consapevole. È una svolta radicale rispetto alla politica dell'assistenzialismo clientelare diretto unicamente ad ammorbare i cittadini, costruendo un sistema di finte garanzie. È una svolta importante rispetto ai paraventi che mistificavano la realtà creando aspettative puntualmente tradite. È una svolta decisiva per liberarci dalle scellerate iniziative che hanno drogato l'economia e imposto a questo Governo interventi per tamponare i disastri del passato recente. Accogliamo con rispetto e con soddisfazione il cambiamento di rotta che riporta il lavoro nella sua veste costituzionale, con progetti seri di politiche attive, che faranno aumentare i tassi di occupazione, con un occhio di riguardo per quella femminile e giovanile, al fine di evitare il collasso del nostro sistema di protezione e sicurezza sociale. Protezione e sicurezza: parole troppo spesso lanciate nelle piazze e molto poco affrontate con un serio approccio dal legislatore. L'Italia, tra *bonus* e regalie, sta scomparendo, signor Presidente: il tasso di natalità ha raggiunto un livello estremamente preoccupante e, se i bambini non nascono, un domani neanche troppo lontano la forza lavoro mancherà; la popolazione al contempo invecchia e ciò significa una spesa pubblica maggiore per garantire la meritata dignità a chi ha lavorato per decenni, a fronte però di minori entrate fiscali. In altre parole, le soluzioni sin qui condotte dalla sinistra in questi anni avrebbero portato l'Italia al collasso. Se manca la manodopera - predica sempre la stessa sinistra di cui sopra - accogliamo diffusamente senza limiti e regole gli immigrati, possibilmente a basso costo, così da far contenta qualche cooperativa amica; che lavorino per mantenere i pensionati italiani: una soluzione anche un po' classista, se me lo permettete. a queste persone non si può solo chiedere lavoro, ma bisogna anche dare la dignità garantita dalle tutele costituzionali: lo stipendio, l'assistenza sanitaria e una casa in cui vivere; cose molto spesso assenti, come viene drammaticamente raccontato dalle cronache recenti. La soluzione immigrazionista della sinistra non può essere, però, la nostra. Noi dobbiamo puntare su politiche che consentano a tutti di programmare un futuro; non possiamo, per carità, classificare persone di serie A e persone di serie B, B, quelle che si utilizzano per propaganda elettorale e si relegano consapevolmente a individui di serie B. Dobbiamo traguardare - e questo è l'impegno concreto del DEF DEF - e consentire alle famiglie di scegliere di avere figli: una scelta consapevole *(Applausi)* e non condizionata dall'ansia di non poter reggere il peso di una famiglia, del lavoro, del costo della vita, degli asili nido - che non ci sono - della babysitter o dei nonni che lavorano fino a settant'anni. Questo significa riportare l'individuo al centro del dibattito e non tradire i nostri avi, che hanno fatto tanto per lasciarci in eredità il diritto di avere una libertà. Questa è una delle priorità del DEF del Governo Meloni: sostegno all'istruzione e all'occupazione femminile, da un lato, e supporto ai nuclei familiari dall'altro, affinché anche avere dei figli possa essere per una donna una scelta di libertà. però, come dicevo, è anche un documento ambizioso, consapevolmente e razionalmente ambizioso, perché, nonostante il contesto geopolitico incerto, con la guerra in corso e le altre situazioni di conflitto che continuano a sorgere in diverse parti del mondo, le politiche monetarie restrittive delle banche centrali globali, il rialzo dei dei tassi di interesse e l'inflazione a livelli altissimi, gli obiettivi fissati sono notevoli. La crescita del PIL - testimoninata anche da chi non è proprio dalla nostra parte, di fronte a una stizzita giornalista che cercava di frenare le parole dell'autorevole amministratore pubblico la riduzione del *deficit* e del rapporto tra debito della pubblica amministrazione e PIL, la decrescita dell'inflazione, il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni, il decremento della pressione fiscale su cittadini e imprese e l'aumento dei tassi di occupazione nelle percentuali previste da questo DEF, infatti, sono indubbiamente obiettivi ambiziosi. L'ambizione è quella giusta, che non spaventa chi lavora indefessamente. Questa è la condizione del nostro Governo e del nostro Presidente del Consiglio. Le riforme indicate nel DEF finalmente riportano al centro le vere necessità economiche e sociali dei cittadini e delle famiglie italiane. pongono un'attenzione speciale su donne, giovani e anziani. *(Applausi)*. Si focalizzano sul lavoro e sui lavoratori di ieri, di oggi e di domani. Hanno uno sguardo particolare sul futuro del nostro Paese, con l'istruzione, la ricerca, l'ammodernamento dell'amministrazione pubblica e la transizione ecologica. Infine, questo DEF è un documento questo DEF è un documento che cambia la narrazione del presente, sottraendolo ai tracciati convenzionali che hanno contraddistinto il sinistro decennio che ci lasciamo alle spalle, perché la differenza con il passato è sensibile: il Governo Meloni è consapevole del momento storico e questa lucidità di pensiero ha consentito di di consegnare un piano concreto, efficace, lungimirante ed economicamente sostenibile, che consentirà di raggiungere gli obiettivi dati in campagna elettorale. Questo è ciò che il Paese si aspetta ed è su queste basi che abbiamo ottenuto la fiducia degli italiani. Abbiamo fatto della coerenza il nostro manifesto e non ci smentiremo.

siamo davanti a un quadro previsionale triennale con un DEF molto realista, basato su stime molto prudenti, che si dovrà realizzare in un insieme di variabili economiche legate ovviamente a un contesto internazionale in continua mutazione. Sappiamo bene di essere usciti da quasi due anni di crisi pandemica e ci siamo trovati con un conflitto armato proprio alle porte dell'Europa, le cui conseguenze hanno inciso a livello globale sui prezzi delle materie prime e dell'energia. Alla conseguente inflazione, causa appunto della crescita del costo dei beni e dei servizi del carrello della spesa, la Banca centrale europea ha risposto con un rialzo dei tassi d'interesse. L'Italia aveva reagito bene alla crisi economica conseguente alla pandemia, riuscendo a cogliere un rimbalzo significativo nel 2021 e nel 2022, dopo la caduta verticale del 2020. Ora il Governo Meloni sta cercando di riportare alla crescita l'economia di un Paese che paga il peso di anni di mancate riforme. ragione il percorso di crescita indicato appare dunque prudente, ma soprattutto realizzabile, alla fine delle tante iniziative di riforma che il Documento indica. ventuno i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, alcuni dei quali hanno già iniziato il loro percorso in Parlamento: dall'adozione di misure per il *made in Italy* a un sistema organico degli incentivi alle imprese, a interventi a sostegno della competitività dei capitali e alle nuove politiche per il lavoro. Gli obiettivi di questo DEF sono quindi chiari e raggiungibili: riformare e semplificare per rimettere in moto l'iniziativa economica privata, privata, utilizzando al meglio le risorse, inserendole in un piano di interventi strutturali per modernizzare l'Italia. In questo contesto, possiamo dire che rientrano uno dei più importanti e puntuali

Era necessaria anche la revisione della spesa pubblica, attraverso il taglio degli sprechi per puntare a servizi migliori, ma soprattutto questo DEF propone una graduale e costante riduzione della pressione fiscale sugli italiani. L'ulteriore riduzione del cuneo fiscale, in parte già iniziata con l'ultima legge di bilancio, arriverà già dal decreto del 1° maggio. Seguirà l'attuazione della delega fiscale, che porterà un'ulteriore riduzione delle tasse, mentre l'opera di semplificazione può aiutare ad avere una macchina pubblica più efficiente. Peraltro, si è già ha cominciato con il nuovo codice degli appalti per la realizzazione delle tante infrastrutture previste dal DEF, che contribuiranno a modernizzare l'intero Paese. Va detto che il DEF dimostra dunque un'attenzione ai conti pubblici e alla spesa ed è pronto a fare i conti con le nuove regole europee del Patto di stabilità che sono state illustrate ieri. ieri. Il Governo deve andare avanti perciò con gli investimenti pubblici, con il sostegno a quelli privati e, nel contempo, con un concreto efficientamento della macchina statale. Se unitamente al livello della produttività privata sale anche quella pubblica, la nostra economia può continuare a creare benessere, affrontando le sfide che ci vengono da un mondo sempre più competitivo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante le migliori intenzioni e i risultati concreti portati a casa dai Governi Conte I e Conte II, che hanno visto la sanità in cima all'agenda politica del nostro Paese, questo Esecutivo ha invertito nuovamente la rotta, relegando il Servizio sanitario nazionale sotto la voce di varie ed eventuali. È doloroso evidenziare che la risposta fornita dal Governo Meloni nel DEF va in direzione diametralmente opposta rispetto alla richiesta avanzata

collocandosi quindi in linea con la media europea dell'8 per cento, il Governo delle destre, il Governo del «siamo pronti», ha previsto una spesa al ribasso del 6,3 per cento per cento nel 2025-2026, senza considerare l'andamento inflazionistico che provocherà un aumento dei prezzi al consumo e quindi anche dell'IVA e delle entrate indirette dello Stato. Vi ricordo che l'IVA, insieme con l'IRAP e con il fondo di perequazione, alimentano il Fondo sanitario nazionale. Questo Governo

nazionale; a diminuire il personale medico e infermieristico nella sanità pubblica; a tagliare ulteriormente i servizi nella sanità, negli ospedali e nei pronto soccorso; soccorso; a privatizzare ulteriormente la sanità. È questo quello che dice il DEF e così lentamente muore il nostro Servizio sanitario nazionale, diventando solo appannaggio di privati e assicurazioni. Questo Governo e queste destre stanno conculcando il nostro modello pubblico di sanità (lo stanno cioè calpestando forzosamente: applichiamo correttamente questo termine) incrementando la sperequazione nell'accesso alle cure con le fasce dei cittadini meno abbienti, che saranno in misura ancora maggiore escluse dal Servizio sanitario nazionale. Il MoVimento 5 Stelle sta tentando sempre, in ogni modo, di lanciare l'allarme contro questa non non più strisciante, ma palese privatizzazione del nostro sistema sanitario. Basti pensare che secondo l'annuario statistico nazionale

per cento di quelle riabilitative. Sempre nel 2021, la spesa sanitaria a carico delle famiglie è stata di ben 36,5 miliardi, con una spesa privata in media di 1.800 euro per nucleo familiare, mentre 4,5 miliardi sono stati a carico delle assicurazioni e dei fondi sanitari, che godono - lo ricordo - di consistenti agevolazioni fiscali che oggi, per circa il 70 per cento, erogano prestazioni già incluse nei LEA, nonostante fossero nati per integrare le prestazioni non offerte dal Servizio sanitario nazionale. Quindi, onorevoli colleghi, privatizzare la sanità vuol dire inevitabilmente portare a un aumento dei costi per i cittadini e soprattutto a un sistema che privilegerà i ricchi e priverà i fragili di cure e di assistenza. *(Applausi)*. È evidente che gli italiani, con un PIL *pro capite* minore, rinunceranno alle cure, così come lo è che le lunghe liste d'attesa, figlie di una sottodotazione del nostro sistema sanitario, costringeranno sempre più i cittadini a rivolgersi alle strutture private, sempre che ne abbiano la possibilità economica. Basti pensare che, sempre nel 2021, i tempi d'attesa per una visita specialistica - questo è l'esame di lealtà che chiedo al Governo - la media è stata di circa cinquantacinque giorni, mentre i tempi d'attesa per un intervento chirurgico sono stati di sessanta. Secondo i recenti dati Istat, che pure qui sono stati pronunciati, indicando l'indice di fiducia dei consumatori - ma io vi chiedo quale sia l'indice di fiducia dei pazienti che aspettano tutti questi giorni - il 7 per cento degli italiani ha già rinunciato alle cure. Così, ogni anno migliaia di pazienti sono costretti ad aspettare mesi per ottenere l'appuntamento per una visita specialistica o un intervento chirurgico, il che impedisce di risolvere tempestivamente le patologie.

nazionale: mancano 60.000 infermieri e 20.000 medici, di cui 10.000 nei reparti ospedalieri e 6.000 nei reparti di medicina generale, 4.500 solo nei pronto soccorso. sarà difficile vincere queste sfide che ci aspettano, con un servizio pubblico sottofinanziato, che ricorre sempre di più a esternalizzazioni, sottopagando il personale, che poi è anche il motivo per cui tanti nostri medici e sanitari sono fuggiti all'estero. Ve lo ricordo: si tratta di 15.000 infermieri e 21.000 medici. La nostra forza politica sta lottando strenuamente per invertire la rotta, presentando...

presentando emendamenti, proposte di legge, interrogazioni e tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione in Parlamento. Abbiamo solamente chiesto ascolto, abbiamo chiesto di rafforzare il sistema pubblico e investire nelle risorse umane e materiali necessarie per garantire un servizio sanitario di qualità e soprattutto equo e uniforme, da Trieste a Lampedusa. Questo DEF non lo dice e non lo consente.

a più riprese nel DEF leggiamo il termine "previsioni di crescita caute". La cautela e la prudenza, in economia come nella vita, sono doti importanti, ma non possono essere confuse con l'immobilismo. La questione vera che emerge nel DEF è non prendersi cura di alcune questioni importanti, per la vita e per il futuro del Paese, vanno affrontate con coraggio e determinazione. Queste previsioni di crescita caute, come le definisce il Governo, in realtà sono nettamente superiori alle previsioni, ad esempio, del Fondo monetario internazionale, che non giustifica, attraverso l'immobilismo del DEF, quella crescita che comunque il Governo prevede. La crescita è determinata dagli investimenti negli elementi strutturali del Paese, per farlo crescere, e se questi mancano, anche se spero non sia così, smentite anche le vostre previsioni di crescita caute e prudenziali. L'unico intervento di politica economica a sostegno della domanda

Per carità, siamo molto lontani dai cinque punti promessi in campagna elettorale, per non parlare dell'inflazione e del recupero dei redditi sull'inflazione, ma è comunque un segnale, che colgo come positivo non può essere uno *spot* annuale. Per il 2024 non si trovano nel DEF quei 10 miliardi indispensabili

se l'anno prossimo i lavoratori si trovassero in una condizione diversa da quella che hanno vissuto quest'anno (parziale, ma significativa). Non si può immaginare che solo per un anno si stia nella sintonia della campagna elettorale e non si preveda, attraverso il DEF, una strategia per l'economia del Paese.

è la mancanza di professionalità adeguate nei Comuni, nelle Regioni e nella pubblica amministrazione. È evidente che, al di là del fatto di denunciare questo aspetto (oggettivo e non in discussione, perché è la fotografia del nostro Paese per quanto riguarda la pubblica amministrazione), ci saremmo aspettati il rinnovo dei contratti pubblici e assunzioni adeguate nella pubblica amministrazione, anche per uscire dal cono della vergogna

questo è insopportabile in un Paese dov'è evidente il danno che si produce non facendo investimenti adeguati nella pubblica amministrazione.

alle proprietà private e alle associazioni delle categorie private che devono rinnovare i loro contratti. Ci sono infatti quasi 7 milioni di lavoratori privati che ancora ancora attendono il rinnovo dei contratti. Per dire questo, il Governo nel DEF deve dare il buon esempio e prevedere le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici. C'è una frase che ricorre nel DEF e che in qualche modo è chiara: il finanziamento degli interventi di politica di bilancio avverrà all'interno del bilancio pubblico. Questo vale per la pubblica amministrazione, per la scuola e per la sanità e "a casa mia" generalmente si traduce in tagli alla pubblica amministrazione (e purtroppo l'elenco va avanti). Arrivo alle politiche attive del lavoro. Anche a questo proposito, da tanti anni leggiamo che ci vogliono interventi importanti e strutturali nelle politiche attive, ma non si stanziano le risorse per farli. Abbiamo l'impressione che l'unica strategia di politiche attive sia quella di tagliare

le linee del suo decreto rispetto alla rivisitazione del reddito di cittadinanza e al lavoro. Questo per quello che leggiamo sulla stampa, perché ad oggi né noi né le parti sociali abbiamo visto nulla, se non qualche bozza continuamente corretta, con cui si rimettono le mani sul tema. Ebbene, invito a non fare l'errore di presentare il 1° maggio qualcosa che ha un significato preciso: tagli al sostegno al reddito, a partire dalla povertà, e allargamento delle maglie sulla precarietà. Sarebbe una provocazione inutile in un Paese che ha già tensioni

tutto il Governo lo sta maturando in splendida solitudine, senza confronto con il Parlamento e con le parti sociali, eppure parliamo di elementi vitali per il futuro del Paese. L'elenco sarebbe lungo,

e una certa passione, della scuola del merito, di cosa significava il termine "merito" e a chi era rivolto, con posizioni anche diverse e articolate, com'è normale in politica, in Assemblea e tra le parti rappresentate. Bene, mettiamoci il cuore in pace: non stiamo più dietro a interpretare il termine "merito", perché sulla scuola nel DEF non c'è nulla *(Applausi)*, quindi la scuola del merito non si farà né premiando gli insegnanti e portandoli a stipendi adeguati a livello europeo, né tantomeno dando possibilità ai nostri giovani e alle nostre giovani. Quanto alla sanità, altri hanno citato, ma è possibile che dopo quello che abbiamo vissuto in questo Paese si abbiano ancora incertezze sulla gestione del PNRR proprio nel settore sanitario e proprio per la sanità territoriale? Per bocca dello stesso ministro Fitto, uno dei motivi che rendono cauti sulla sanità territoriale è la mancanza di personale. Bene, allora si deve provvedere e immaginare da subito di impostare un piano di assunzioni nella sanità.

credo che oggi in quest'Aula sia avvenuto un fatto storico, perché anche il presidente Monti ha avuto parole di elogio e ha dato il benestare a questo DEF. Possiamo dire che ormai è certificato, perché ce lo dice anche il presidente Monti, che questo è il DEF dell'austerità, del taglio alle spese e dei sacrifici. Ormai possiamo mettere su questo DEF il sigillo di garanzia, il timbro del presidente Monti, così siamo almeno sicuri di cosa stiamo parlando. consentitemi di chiedervi: cosa state raccontando ai vostri elettori oggi, dopo tutte le promesse che avete fatto in campagna elettorale? Cosa state raccontando agli imprenditori, alle famiglie, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai medici e agli operatori dei pronto soccorso? Cosa state andando a raccontare oggi con questo DEF? Con quale faccia vi state presentando oggi ai vostri elettori, dopo tutto quello che avete promesso in campagna elettorale? Io l'ho letto: è un DEF - sembra veramente che siate ancora in campagna elettorale - di buoni auspici e promesse; non ci sono misure concrete a sostegno di quello che sta succedendo. Forse non vi siete resi conto che l'inflazione ha completamente distrutto i salari da fame che abbiamo in questo Paese, che non crescono da trent'anni. Voi non dovete solo considerare quello che va nelle tasche dei cittadini con il loro stipendio, ma i costi che sono arrivati alle stelle: il carrello della spesa, i prezzi energetici e la sanità privata che state sostenendo, per cui oggi un cittadino per curarsi dovrà trovare anche i soldi per pagare le visite specialistiche a pagamento. Capite che non c'è solo una forma di salario diretto, ma anche indiretto, che è costituito dall'aumento dei costi che le famiglie stanno sostenendo in questi mesi, da quando siete al Governo? Siamo assolutamente insufficienti su tutti i fronti, soprattutto su quello dei salari. Serve assolutamente un adeguamento dei salari a quanto accaduto negli ultimi mesi. negli ultimi mesi. Da un lato, sentivo qualcuno dire che non ci sono i fondi, poi dall'altro lato ci dicono che il presidente Conte ha preso troppi soldi per il PNRR. PNRR. Dovete anche fare pace con voi stessi, perché se da un lato non ci sono i soldi per il superbonus e per le misure espansionistiche e dall'altro

sull'efficientamento energetico delle case, anche con la misura che avete modificato, con un superbonus al 90 per cento. Cerchiamo misure, come il superbonus, che ha creato posti di lavoro, PIL, economia e crescita; cerchiamo di utilizzare almeno i fondi che non riuscite a utilizzare. Prima si diceva Prima si diceva che lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti: guardate che i nostri figli e i nostri nipoti ci chiedono tutt'altro; ci chiedono misure coraggiose, spaventati dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli sconvolgimenti che ci potranno essere nei prossimi anni, non ci chiedono misure di di prudenza. Non ci possiamo assolutamente rassegnare all'atteggiamento attendista che state avendo. se abbiamo soldi in più nel PNRR, cerchiamo di spostarli sulle case *green*, cerchiamo di capire che se stiamo demolendo la sanità pubblica dobbiamo ragionare anche in termini di prevenzione delle malattie. Guardate che quando si parla di mobilità elettrica, anche qui fortemente danneggiata, significa eliminare dalle nostre città l'inquinamento che causa tantissime malattie. Questo non è da sottovalutare, perché è vero il fatto che il combustibile viene atomizzato nella camera di combustione, producono meno inquinamento, ma si tratta di un inquinamento molto più pericoloso, perché producono molto più PM 2,5, quindi è un inquinamento che penetra nei polmoni e nei sistemi cardiocircolatori delle persone e causa le malattie che stiamo osservando oggi. Abbiamo tantissimi tumori ai polmoni nei non fumatori e leucemie:

nelle nostre città, proprio in un'ottica di prevenzione. Non possiamo continuare ad avere macchine inquinanti vicino alle scuole, dobbiamo almeno eliminarle. *(Applausi)*. Non potete essere d'accordo con l'Europa quando vi chiede austerità e poi contro l'Europa quando ci chiede case *green* e mobilità Non potete essere d'accordo su quello che non conviene al nostro Paese e poi essere d'accordo su ciò che causa danni. danni. Dovete cambiare registro, anche perché nell'allegato 4 - non so se ve ne siete accorti - quando parlate di misure a sostegno degli obiettivi europei sul Fit for 55, avete lasciato ancora il superbonus che avete demolito. Avete inserito come misure prioritarie superbonus e comunità energetiche, quando i decreti attuativi sulle comunità energetiche mancano da un anno. *(Applausi)*. Avete almeno letto cosa avete scritto nell'allegato 4 al DEF? State puntando sui nostri cavalli di battaglia dopo che li avete distrutti e quando mancano i decreti attuativi da sette mesi. Cosa andate a scrivere in questo DEF?

un aiuto a spendere meglio i soldi del PNRR, per avere investimenti produttivi. Se non capite che spendiamo 40-50 miliardi l'anno per comprare fonti fossili dall'estero

non dando contentini. Dobbiamo mettere questo Paese in condizione di sfruttare le risorse interne, che sono altamente convenienti dal punto di vista economico, solarizzando tutti i tetti e rendendo quell'energia condivisa, stabile e a basso prezzo. Questo è quello che ci chiedono i nostri giovani,

e interventi strutturali per rendere questo Paese sostenibile e soprattutto vivibile nei prossimi anni.

il Documento di economia e finanza 2023 è un atto fondamentale per il Governo

economico è sicuramente in miglioramento, ma sappiamo anche che le condizioni geopolitiche internazionali e il perdurare del conflitto russo-ucraino russo-ucraino non avvantaggiano la situazione economica che stiamo vivendo. Pensiamo solo al rialzo dei tassi di interesse e al drenaggio di liquidità operato dalle banche centrali che hanno fatto affiorare sacche di criticità preoccupanti nel sistema bancario internazionale.

Ci sono indicatori che ci danno una lieve ripresa della crescita economica, confermata anche dalle indagini presso le imprese italiane,

prima di tutto alla sanità). È stato detto più volte che in questo Documento non c'è nulla di serio sul tema della sanità

no? Sappiamo che non ratificare il MES - come ci è stato detto anche ieri dall'Europa - significa bloccare di fatto alcune riforme prioritarie che servirebbero al nostro Paese. Non sto qui ad elencare tutti i motivi per cui in questo momento sarebbe necessario investire risorse economiche proprio sulla sanità. Cito soltanto per titoli alcune questioni che sono state riprese anche da altre colleghe e da colleghi che mi hanno preceduto: il tema della carenza del personale medico e infermieristico le liste d'attesa, su cui, per esempio, Italia Viva e Azione già tempo fa avevano lasciato proprio al presidente Meloni importanti proposte per migliorare il sistema sociosanitario italiano. Questo è sotto gli occhi di tutti. Potete dire ciò che volete, che non accettate il MES e che non volete fare altri investimenti, ma, se parlate e vi connettete con gli italiani, con i cittadini, con le comunità e con i sindaci, scoprirete che la realtà è un'altra, perché ci sono problemi enormi sul sistema sanitario anche in quelle Regioni dove la sanità è sicuramente più solida rispetto ad altre. Questo accentuerà ancora di più le diseguaglianze tra aree geografiche, Nord, Centro e Sud. Non lo diciamo perché vogliamo essere contro, ma perché vogliamo venirvi incontro rispetto ad alcuni temi che consideriamo prioritari. Il Sistema sanitario nazionale deve garantire garantire livelli essenziali di assistenza (LEA) per tutti, e oggi sappiamo che ancora non è così, nonostante le raccomandazioni e anche

che servono le risorse importanti del MES. Altro tema che mi sta a cuore, che è un pilastro e un'altra gamba del sistema di *welfare* del sistema sanitario, è lo sport. Ne abbiamo parlato tanto, anche in queste Aule, abbiamo un Ministro competente in questo senso. Anche oggi in 1a Commissione si è votato sull'ingresso dello sport in Costituzione, aggiungendo un comma all'articolo 33 della Carta, quindi all'interno del diritto all'istruzione, facendo in modo che lo sport possa diventare un diritto di tutti e per tutti, e accanto all'articolo 32 della Costituzione, quindi il diritto alla salute.

e che lo sport non è ancora visto come un investimento sulla salute e sulla prevenzione, a cominciare proprio dai bambini. Questo avrebbe un grande impatto significativo benefico sull'aspetto sociosanitario. Il ministro Abodi, nei giorni corsi, rispondendo anche a una nostra interrogazione, ha confermato che la riforma dello sport entrerà in vigore il 1° luglio 2023.

che ci ha convinto su alcuni aspetti, ma ha già messo le mani avanti rispetto ad altri progetti che invece non vedranno la luce entro il 2026 - dobbiamo essere seri, dobbiamo essere seri, responsabili e soprattutto onesti verso gli italiani, raccontando la verità. Non si può pensare di essere sempre in campagna elettorale:

tuttavia dover constatare ancora una volta oggi che, di fronte a un Documento così importante, purtroppo non abbiamo le aspettative di crescita e gli obiettivi che pensavamo invece ci fossero dopo un Governo importante come quello come quello Draghi, che vi ha lasciato sicuramente una situazione migliore di quella passata. Ebbene, forse qualche passo in avanti in più lo potevate fare. **Saluto

mi concederete di iniziare il mio intervento - e sono molto emozionata per questo - dedicando un pensiero sentito e profondamente commosso alla dottoressa Barbara Capovani e alla sua famiglia. Barbara era una bravissima psichiatra della mia città, Pisa, ed è morta per mano di un suo paziente in una dinamica che genera rabbia e dolore. Non sono ore facili quelle che sta vivendo la nostra comunità e non è facile per me - ve lo confesso - dover pronunciare queste parole.

Quasi per uno scherzo del destino nel mio intervento sono chiamata ad affrontare il tema di ciò che lo Stato prevede di fare nel DEF per sostenere il sistema sanitario nazionale e a trattare, tra le altre, le problematiche che affliggono il personale sanitario (medici, infermieri e operatori sociosanitari). Lo hanno già detto le mie colleghe Furlan e Camusso, ma lasciatemi dire, senza troppi giri di parole, che purtroppo quanto viene previsto mi pare del tutto insufficiente e vengo alle ragioni di tale giudizio. Su tutte c'è il fatto che questo DEF, il primo del Governo Meloni, si caratterizza per una preoccupante assenza di visione, di strategie e, soprattutto, di risorse. Le risorse, appunto: è da qui che vorrei partire per provare a spiegare le ragioni della nostra preoccupazione. Nel triennio 2024-2026, a fronte di una crescita media annua del PIL nominale del 3,6 per cento, questo DEF nel 2023 stima quella della spesa sanitaria allo 0,6

per poi risalire nel 2025 a 135 milioni (+1,7 per cento) e a 138 milioni nel 2026. Sono numeri che prevedono un aumento medio così misero da non essere in grado nemmeno di coprire l'aumento dei prezzi dovuto all'inflazione. Ricordo che secondo l'OCSE il limite di sostenibilità di ogni sistema sanitario nazionale è il 6,6 per Non si pensi che il Sistema possa reggere semplicemente facendo crescere il secondo pilastro, quello della sanità privata. Del resto, sembra questa la strategia di questa maggioranza che si riscontra, ad esempio, da quel che succede in Veneto e che ho letto in un'inchiesta pubblicata la scorsa settimana sul La sanità privata è cresciuta in Veneto del 434 per cento in undici anni, ma - come dicono tutti gli esperti - mettere in competizione la sanità pubblica con quella privata ha solo come risultato di far soccombere la prima. Sono mesi che proviamo a chiedere a gran voce un'attenzione sul tema della sanità pubblica. La risposta del Governo è in questo testo che stiamo discutendo e non considera la sanità una priorità perché continua a non mettere al centro la salute delle cittadine e dei cittadini di questo Paese. Lo dico non solo con grande rammarico, ma anche con una profonda perché le risposte che non siamo in grado di costruire in queste Aule hanno un impatto enorme sulla vita dei cittadini, a partire da quella del personale sanitario, su cui - me lo concederete - vorrei fare un piccolo *focus*. In tanti avrete letto i dati OCSE e il rapporto Crea che ci dicono che mancano circa 150.000 infermieri e non i 65.000 che vengono riportati nella NADEF. Ancora mancano circa 30.000 medici, di cui 4.500 nei pronto soccorso, 10.000 nei reparti ospedalieri e 6.000 medici di medicina generale. Se poi si considerano i pensionamenti previsti nei prossimi anni, si arriva a cifre da capogiro. Per amore di verità, dobbiamo dire che i tetti di spesa per il personale sanitario li ha decisi per la prima volta il Governo Berlusconi nel 2011.

Ecco, si sarebbe dovuto continuare su questo binario e invece questo Governo vuol imprimere un'inversione di marcia, girandosi totalmente dall'altro lato.

dirigenti sanitari, è insoddisfatta delle condizioni del proprio lavoro, perché i medici sono pochi e mal retribuiti. C'è poi il capitolo PNRR: un'occasione unica per il nostro Paese, che il Governo sembra voler gettare alle ortiche. In questo DEF ci sono riferimenti astratti ed evasivi che denotano tutta l'inadeguatezza del Governo, perché sembrano arrendersi all'idea che l'attuazione della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza non sia alla nostra portata. Ciò sembra confermato dall'informativa resa ieri in quest'Aula dal ministro Fitto: non un accenno alla Missione 6, e questo sarebbe di una gravità inaudita, perché noi, con quel pezzo di missione, possiamo garantire ai cittadini la realizzazione di 1.350 case di comunità, 400 ospedali di comunità, 600 centrali operative territoriali e lo sviluppo della telemedicina in grado di assistere 800.000 persone con più di a casa propria. Per non parlare del tema della digitalizzazione, su cui le risorse investite sono importanti e su cui credo il Governo dovrebbe porre la massima attenzione. Ecco, questi investimenti avrebbero un impatto positivo proprio sulla spesa corrente su almeno tre fronti: la riduzione dei ricoveri non necessari in caso di patologie croniche, la diminuzione del ricorso inappropriato ai pronto soccorso, la riduzione della spesa per alcune tipologie di farmaci ad alto rischio di inappropriatezza. Per questo nei prossimi giorni chiederemo al ministro Schillaci un confronto di merito sullo stato di attuazione della Missione 6 per superare eventuali ritardi e inadempienze. Capiamoci: qui tutti noi facciamo il tifo per l'Italia e ci auguriamo che il Governo sia in grado di rispondere agli impegni che il nostro Paese ha assunto. E lo facciamo, signor Presidente, perché crediamo che sulla salute delle persone, sul loro futuro sulla loro dignità non ci sia dibattito politico che tenga. Ho esordito ricordando la memoria di Barbara e l'enorme sacrificio che quotidianamente affrontano i nostri operatori sanitari. Signor Presidente, onorevoli

In questo DEF - ahinoi - di impegno se ne vede veramente poco. Anche per questo continueremo la nostra battaglia a difesa della sanità pubblica, in queste Aule, nelle nostre città e nelle nostre piazze. *(Applausi)*.

prudente, ma realistico, di questo DEF, che è stato anche autorevolmente riconosciuto dal presidente Monti. Solo che essere realisticamente prudenti non significa rinunciare ai programmi che si vogliono realizzare.

ogni anno una maggioranza differente. Abbiamo una maggioranza, perché il popolo è con noi e ci ha votato, quindi ragioniamo su questa prospettiva. Chiaramente

tanti fattori legati al caro energia, che per fortuna si sta riducendo, ma sui quali - nessuno l'ha citato - proprio il Governo Meloni, in sede di finanziaria per il 2023, aveva provveduto a porre risorse importanti, per mitigare l'effetto sulle famiglie e sulle imprese, addirittura con un una previsione che si è rivelata per fortuna eccessiva. Quelle stesse risorse sono state riprogrammate per ulteriori aiuti,

cui il Governo Meloni vuole privatizzare la sanità e abbandonare la sanità e il Servizio sanitario nazionale. Vorrei sapere in quale rigo del DEF è scritto che vogliamo abiurare a una missione principale prevista dalla Costituzione, cioè quella di tutelare la salute dei cittadini. Non lo vedo, non l'ho trovato, onestamente. Ho trovato invece una visione realistica, che cerca di aumentare le risorse, alle condizioni finanziarie attuali, per il Servizio sanitario nazionale, in una prospettiva prudente,

utilizzare i soldi del PNRR per la salute. Non l'ho visto scritto, anzi si parla del fascicolo elettronico, di case e di ospedali di comunità (si parla di attuare questa parte). Certamente, dobbiamo trovare anche il personale per riempire poi le case di comunità. Lo sappiamo, che siamo al Governo da sei mesi. C'è stata una maggioranza diversa per dieci anni: gli autorevoli esponenti del PD cosa hanno fatto per dieci anni al Governo? ma i tetti per personale e il problema della mancanza dei medici c'erano prima? Penso di sì. Poi ce ne siamo dovuti accorgere con la pandemia, che è stato un evento devastante, di cui ancora scontiamo gli effetti. In questo contesto, il collega Scurria prima diceva che abbiamo smentito i profeti di sventura, che pensavano che l'arrivo di Giorgia Meloni e della destra al Governo portasse l'arrivo delle cavallette o non si sa quali cataclismi epocali. No: ha portato semplicemente una forza politica, insieme a tutto il centrodestra, che con sano realismo, contrapposto all'ideologismo onirico di chi ha pensato sempre che le case degli altri si potessero ristrutturare gratuitamente a spese della comunità, affronta gli argomenti passo passo,

per la Nazione, chiede rispetto per l'Italia e non si abbassa a dire semplicemente che ce l'ha detto l'Europa, ma ha obiettivi importanti. Ha l'obiettivo di creare sviluppo occupandosi di natalità, di crisi demografica

in un meccanismo che, invece di creare inflazione, cerca di andare incontro alla necessità di recuperare potere d'acquisto da parte dei salari. Tutto questo lo faremo passo passo, bisogna che ci si rassegni;

ma soprattutto perché siamo convintamente italiani e vogliamo far vincere la nostra squadra, la squadra dell'Italia. Altri invece non sembrano far altro che gufare affinché questa squadra perda.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare una cosa: fondamentalmente penso - come ho già avuto modo di dire nelle audizioni in Commissione che questo DEF non abbia alcuna visione. La linea che la maggioranza tiene è quella della prudenza. Giusto, bisogna essere prudenti e non metto in discussione la prudenza, ma non ha una visione, perché credo che il Documento

Questa mattina noi di Verdi e Sinistra in molte città stiamo distribuendo volantini sulla nostra opinione sulla questione della sanità e riscontriamo ovviamente nei cittadini e nelle cittadine un consenso rispetto a quanto portiamo avanti. Qual è la situazione? È stato detto anche prima che non è vero che c'è una riduzione della spesa. Il documento della Banca d'Italia, presentato in audizione la settimana scorsa - quindi non l'abbiamo scritto noi - dice che si passa dal 6,9 al 6,2

che finanzia la sanità pubblica. Siamo ora in una situazione in cui siamo usciti dalla pandemia.

non per il personale. È vero che è scritto in questo modo, ma, se si vuol fare la sanità territoriale, bisogna anche prendere del personale e quindi individuare uomini e donne che riempiano le case di comunità, altrimenti è un po' complicato pensare di fare sanità territoriale.

Credo che dobbiamo fare una grande riflessione e questo vale per tutti. La sanità regionalizzata, così com'è stata fatta in questi anni, e addirittura adesso con l'autonomia differenziata, ha senso?

di vista occupazionale, anche se purtroppo precario, perché si ragiona in emergenza: ha dato un'occupazione di circa 900.000 posti, ma precari. Il problema è che si è cancellata questa norma e non si fa nulla

2023, si compone di tre sezioni: la prima, relativa al programma di stabilità; la seconda, relativa alle analisi e tendenze della finanza pubblica; la terza, relativa al Programma nazionale di riforma. In questo mio intervento, Presidente, mi occuperò soltanto del settore giustizia, nel quale - come credo sia noto a tutti in quest'Aula - si articola la maggior parte del mio impegno parlamentare. Il DEF 2023, nella prima sezione, espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2022 e le previsioni tendenziali e programmatiche per il 2023 e per il triennio successivo. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica e fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione del documento stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto delle politiche economiche prospettate all'interno del Programma di stabilità e del Piano nazionale delle riforme, che saranno successivamente definite nella Nota di aggiornamento e quindi adottate con la prossima legge di bilancio. Quanto ai disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, il Documento menziona, per quanto riguarda la giustizia, i seguenti disegni di legge concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; la rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e la ridefinizione dei ruoli professionali anche con riferimento al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; gli interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena. Con riferimento al riordino della geografia giudiziaria, qualche perplessità si desta si desta con riferimento all'ipotizzata riapertura dei cosiddetti tribunalini, nei quali a parità di organico, con tutta evidenza, non potranno essere garantiti né specializzazione, né efficienza, né tantomeno qualità di giurisdizione. Con riferimento alla II Sezione, recante analisi e tendenze della finanza pubblica, vengono in rilievo in particolare le tabelle di dettaglio concernenti l'analisi economica dei pagamenti effettuati nel triennio 2020-2022. Nella III Sezione, recante il Programma nazionale di riforma, il Governo presenta una stima aggiornata dell'impatto macroeconomico del PNRR che si basa sulle spese effettuate nel triennio 2020-2022. In particolare, il Programma nazionale di riforma reca un aggiornamento della valutazione d'impatto macroeconomico delle riforme, con specifico riguardo a quelle del settore della giustizia che comporteranno un incremento di 0,4 punti percentuali del PIL nel 2006, di 0,6 0,6 punti nel 2030 e di uno 0,7 per cento nel lungo periodo. Sono dati che personalmente reputo significativi. Con riferimento al settore di competenza, il DEF evidenzia lo stato di avanzamento della riforma del sistema giudiziario, che rappresenta una delle sfide di maggior rilievo che l'Italia si è impegnata ad affrontare nell'ambito del PNRR. Al riguardo, il Documento evidenzia come proprio il Programma nazionale di riforma (PNR), al fine di migliorare la celerità e l'efficienza del sistema giudiziario, abbia stanziato circa 3 miliardi di investimenti che spaziano dal rafforzamento del capitale umano al funzionamento dell'ufficio per il processo alla transizione digitale del sistema giudiziario, fino all'efficientamento del patrimonio immobiliare. Tali interventi devono affiancarsi alle riforme strutturali previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'obiettivo principale per il settore giustizia è rappresentato dall'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari in Italia. Nel 2022 sono state già adottate le seguenti riforme: la riforma del processo civile, la riforma del processo penale, la riforma delle procedure di insolvenza e la riforma della giustizia tributaria. Più nel dettaglio, Presidente, la riforma del processo civile ha avuto l'obiettivo di realizzare una riforma organica e di riassetto strutturale, volta ad accelerare il processo di cognizione, il processo di esecuzione, i procedimenti speciali e a incentivare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. La maggior parte delle disposizioni contenute nella riforma sono divenute efficaci a decorrere dal 28 febbraio scorso, come stabilito nell'ultima legge di bilancio. Conseguentemente, l'articolo 35 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha disposto l'anticipazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti al 1° marzo 2023, ivi compresi i provvedimenti e i verbali di udienza dei magistrati anche ai procedimenti pendenti alla medesima data. La riforma del processo penale, entrata in vigore il 30 gennaio 2022, è stata invece diretta a realizzare l'obiettivo di ridurre i tempi di trattazione del 25 per cento rispetto al 2019, attraverso interventi di razionalizzazione, deflazione e accelerazione dei provvedimenti che incidono su diversi profili. La riforma delle procedure d'insolvenza, considerata prioritaria nell'ambito del PNR, è volta a offrire agli imprenditori strumenti più efficaci per sanare le situazioni di squilibrio economico patrimoniale che appaiono reversibili, quali ad esempio la composizione negoziata delle crisi d'impresa e i meccanismi di allerta precoce. Con decreto legislativo n. 83 del 2022, il Governo ha infatti fatto confluire nel codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza le disposizioni sulla composizione negoziata della crisi introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021. Il codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022, in anticipo rispetto al traguardo previsto nel PNR, fissato al 31 dicembre 2022. La riforma della giustizia tributaria, che è stata sancita con legge n. 130 del 2022, ha l'obiettivo di rendere più efficiente il processo e di ridurre l'elevato numero di ricorsi per Cassazione. Sono previste misure ordinamentali e processuali con finalità deflattive e di accelerazione dei giudizi, tra cui la professionalizzazione dei giudici, il potenziamento delle strutture amministrative e il rafforzamento dell'autonomia dell'organo di autogoverno. La legge è entrata in vigore il 16 settembre 2022, rispettando le previste tempistiche del PNR, che richiedevano una riforma delle commissioni tributarie entro il 31 dicembre 2022. Qualche problema si sta riscontrando nel reclutamento dei magistrati togati professionali. A tale proposito sarà necessario, in tempi brevi, qualche ulteriore ritocco normativo per garantire che gli obiettivi della riforma siano ottenuti effettivamente. Per quanto riguarda le riforme del processo civile, del processo penale e delle procedure d'insolvenza, si rileva che, nel corso del 2023, si prevede l'adozione di decreti legislativi correttivi e di atti attuativi. Nel DEF si dà conto di come gli interventi realizzati negli ultimi anni abbiano cominciato a produrre effetti significativi sulla durata dei processi civili e penali, e di questo, Presidente, non possiamo che compiacerci: vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta. In particolare, nel periodo 1° ottobre 2021-30 settembre 2022 la durata dei processi civili è diminuita di circa il 6 per cento presso i tribunali e le corti d'appello e del 26 per cento presso la Corte di cassazione e la durata dei processi penali è diminuita del 7,5

Si tratta quindi di attuare ulteriormente le riforme che stanno dando i loro frutti. Tempi ragionevoli dei processi civile, penale e tributario ci avvicinano a *standard* europei. In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le corti d'appello. Per quanto riguarda i profili organizzativi, il Documento dà conto del reclutamento straordinario al 31 dicembre 2023 di 7.830 funzionari per l'ufficio del processo, nonché del reclutamento - sempre al 31 gennaio 2023 - di 3.406 figure professionali giuridico-amministrative e tecniche per il supporto delle cancellerie e degli interventi di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria. Com'è noto, il il personale amministrativo è fondamentale per il buon andamento degli uffici giudiziari ed è molto positivo che l'attività di reclutamento proseguirà anche nel corso del 2023. Il Governo nel DEF ribadisce inoltre l'impegno ad adottare diversi strumenti per la digitalizzazione del sistema giudiziario. Ricordo al riguardo che, tra gli impegni previsti dal PNRR per il 2023, vi sono la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti, il processo civile telematico, la digitalizzazione dei procedimenti penali, la creazione di una banca dati delle decisioni civili gratuita e pienamente accessibile e consultabile. Nell'ambito degli obblighi internazionali e delle riforme ordinamentali da attuare, nel DEF si dà infine conto dell'approvazione - da parte del Consiglio dei ministri - del disegno di legge sul codice dei crimini internazionali, nonché dell'adozione di provvedimenti volti ad adempiere a obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea in materia di operazioni societarie transfrontaliere, *class action*, contrasto alla diffusione di materiale terroristico *online*. Il documento sottolinea infine che sono in corso di elaborazione di elaborazione disegni di legge in materia di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, di criminalità minorile e di disciplina delle intercettazioni e in materia civile è allo studio un intervento di efficientamento dei relativi crediti. A questo punto, non posso che applaudire le intenzioni del Governo e manifestare l'incoraggiamento mio personale e dell'intero Gruppo Forza Italia al Governo stesso. Risultano altresì allo studio i decreti attuativi della legge delega della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore edilizia carceraria. Come Forza Italia, Presidente, non possiamo che condividere l'operato del Governo, come dicevo poc'anzi, sui temi della giustizia, e fin d'ora confermiamo il nostro sostegno al lavoro e all'impegno del ministro Carlo Nordio. *(Applausi)*.

Rivediamo un *replay* - anche mal fatto - delle politiche del 2008 post-crisi, che hanno portato il Paese quasi al tracollo, con i fatti che tutti ricordiamo. Vediamo una contrazione della spesa, nessuna politica per gli investimenti, nessuna politica industriale, nessuna spinta al motore Paese: solo contrazioni sul fondo sanitario nazionale, che apparentemente cresce come cifra nominale,

dobbiamo tenere il passo, per cui deve crescere la spesa, anche quella riferita alla nostra sanità. Allo stesso modo, dovrebbe crescere la spesa per le retribuzioni dei dipendenti pubblici, ma anche di questa nel DEF non c'è traccia. I contratti sono scaduti. Nel DEF c'è il rinnovo contrattuale 2019-2021: ma, signori, siamo nel 2023. Dove sono le risorse per il rinnovo 2022-2024? Assenti anche queste dal DEF, così com'è assente una politica di sostegno ai salari. Vediamo che si cerca timidamente di difendere le retribuzioni attraverso un fantomatico taglio del cuneo fiscale, che, se fate i conti sui potenziali 19 milioni di lavoratori che potranno beneficiarne, fa l'astronomica cifra di poco meno di 20 euro al mese: non ci si paga neanche una pizza il sabato sera. E questo per i lavoratori che ne potranno beneficiare, perché poi vi dimenticate sempre i *working poor*, gli stessi che purtroppo beneficiano del reddito di cittadinanza come integrazione al reddito, perché non arrivano neanche

stabilisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza

le entrate pubbliche per far pagare il conto dell'inflazione, invece che alle imprese, che aumentano i profitti, allo Stato, alla spesa sociale e agli interventi pubblici. Dove andiamo in questo modo? Dove volete portare il Paese? Di nuovo sull'orlo del baratro? Parliamo di un problema che toccate nel DEF, quello della denatalità, perché siete voi che scrivete che con questo ritmo tra qualche anno nel il *deficit* e il debito pubblico saliranno alle stelle. E quali sono gli interventi? Nessuno, perché la denatalità non si combatte con misure *spot*, come quelle che voi proponete. La denatalità si combatte dando ai giovani, a chi vuole costruire una famiglia, una visione per il futuro, un'aspettativa e una speranza di miglioramento, mentre l'ascensore sociale nel nostro Paese è bloccato. Da alcuni anni nel nostro Paese le nuove generazioni stanno peggio di quelle che le hanno precedute e in questo modo il problema della denatalità non può che peggiorare. I nostri giovani devono avere un lavoro stabile, perché non è con un lavoro "figo", come ha detto uno dei vostri Ministri,

Siamo in Aula: un lavoro "bello". ogni caso, il mutuo non viene concesso con un lavoro precario a sei mesi. C'è bisogno di contratti a tempo indeterminato perché una banca consenta di acquistare una casa.

se perdi il lavoro o vuoi occuparti dei tuoi figli e il lavoro non te lo consente, soprattutto quando sei un libero professionista, poi hai estrema difficoltà a ritrovarlo. Nel PNRR c'era una clausola che prevedeva la parità di genere nell'affidamento dei lavori, ma sparisce nel codice degli appalti, svanendo nel nulla. È così che difendete il lavoro femminile? Posso capire che in alcuni settori potesse essere di reale ostacolo, ma allora andava circoscritta, senza fare di tutta l'erba un fascio; invece, come al solito, buttate il bambino con l'acqua sporca. In conclusione, Presidente, ci aspettavamo di più dal Governo che ha annunciato di essere pronto a guidare questo Paese. Ci aspettavamo una visione, ma non solo noi, persino Confindustria si aspettava qualcosa di più. Non avete fatto nemmeno le politiche per i vostri potenziali elettori. Non c'è niente. Ci auguriamo una possente inversione di tendenza nelle prossime misure, perché così il baratro è sempre più vicino.

consumare tutto il poco tempo che si ha a disposizione per correggere alcune lievi imprecisioni che si sono sentite dire dai colleghi in diversi punti.

doverosa. C'è qualcuno però che dovrebbe fare pace con il cervello, perché da una parte dice che bisogna giustamente alzare gli stipendi e quindi fare misure inflazionistiche e, dall'altra parte, si duole del fatto che, guarda

tal proposito, già che parliamo d'inflazione, è forse il momento di fare una discussione o una riflessione che dovrebbe riguardare tutti, perché tutti sappiamo quanto poco potere abbiamo in quest'Aula. Quando arriva la legge di bilancio, la quota riservata all'analisi del Senato è sempre pari a pochi milioni di euro. Dall'altra parte, invece, il bilancio dello Stato è impattato da variabili - l'inflazione è una di queste - che si spostano per miliardi o per decine di miliardi di euro. Ebbene, direi che l'inflazione è proprio uno di quei fattori. Vediamo un Vediamo un tentativo neanche troppo nascosto di accerchiamento, in questi giorni, da parte di alcuni poteri fortissimi nei confronti del nostro Governo: avete visto in sequenza muoversi Goldman Sachs, che dice del nostro debito "Oddio che brutto, signora mia!", e abbiamo visto le famigerate agenzie di *rating*, che erano state protagoniste di altre stagioni non particolarmente brillanti della nostra storia recente, già subito iniziare a muoversi, immaginare il *downgrade* e di declassare il nostro debito. Tutto questo

sommessamente ricordare che, nonostante tutti questi tentativi sempre più sguaiati e nonostante non vi sia più un centesimo di acquisto da parte della Banca centrale del nostro debito, lo *spread* è tranquillamente a quota 180 e, già che ci siamo, vorrei ricordare com'era lo *spread* con altri fenomeni al Governo, oltretutto, nella maggior parte dei casi, coadiuvati da forti acquisti da parte della Banca centrale. Ricordo lo *spread* a 300 del luglio 2013, con Letta Presidente

A tal proposito, ho osservato con un certo sorriso i richiami neanche tanto velati al MES: mi raccomando, prendete il MES, altrimenti non va bene. Mi rivolgo alla senatrice Sbrollini, che non si sa come mai insista a pensare a questo famoso MES sanitario, che lei e il suo partito delineano

quando sono arrivato, nel 2018, quella tabella l'ho vista. Forse è il caso di ricordargli che è vero che, se domani moriamo tutti, il debito rimane lì, le persone si dimezzano e il debito *pro capite* aumenta; la stessa roba, se si raddoppiano e tutti lavoriamo come stiamo lavorando adesso.

Per il resto, chiudo ricordando che in questo momento c'è un'importante negoziazione sul Patto di stabilità. Quando si dice che noi vogliamo che gli investimenti rimangono fuori dai conti europei su cui si calcoleranno

senza nessun motivo (perché abbiamo visto che l'austerità fa danni al nostro Paese), guardate che questo lavoro diventerà poco piacevole sia per noi in maggioranza sia per voi all'opposizione. vorremmo che essere eurocritici tornasse di moda. Avviso quindi subito che è il caso che si parli con una voce sola, perché queste regole, così come si prospettano, rischiano di non essere particolarmente positive per l'Italia.

intanto tengo a precisare, come ha ricordato anche il presidente Monti, che siamo di fronte a un passaggio cruciale

perché discutere del più importante documento di politica economica e finanziaria in capo al Parlamento - ovviamente mi riferisco al Documento di economia e finanza - senza la presenza del Ministro preclude a quest'Assemblea la possibilità di avere la sua replica in un dibattito che ritengo cruciale e indispensabile per lo sviluppo economico e sociale di questo Paese. C'è una maggioranza politica legittimata dal voto dei cittadini, alla quale è chiesto di governare i cambiamenti di dare una visione e un indirizzo di politica economica e sociale importante in capo ai Governi, alla maggioranza e al Parlamento. Non è consentito, a mio avviso, continuare una campagna elettorale permanente: negli interventi dei colleghi della maggioranza, riscontro una propensione a configurare una campagna elettorale permanente e a richiamare le responsabilità del passato, quando di fronte a noi ci sono sfide e trasformazioni inedite alle quali questa maggioranza, a mio e a nostro avviso, dà e ha dato fin qui soluzioni inadeguate, precarie e ingiuste. Voglio spiegare perché non ci fidiamo dell'abito configurato su misura più per rassicurare i mercati che per affrontare i problemi reali delle famiglie e delle imprese italiane. Non ci fidiamo perché i primi provvedimenti di questo Governo sono stati tutti orientati e finalizzati a un dibattito che va in senso opposto al bisogno e alle esigenze del Paese. Il Partito Democratico lo incontrerete lì, se la vostra narrazione propagandistica elettorale si trasformerà in un confronto reale sulle dinamiche vere dell'economia e della società italiana. Voglio fare un esempio per tutti. Di fronte a una scelta che noi abbiamo sempre proposto e condiviso, poiché la priorità numero uno in questo Paese è ridurre la pressione fiscale sul lavoro per aumentare i salari, aggiungiamo che servirebbe una battaglia di tutti per contrastare la precarietà. *(Applausi)*. Nella precarietà, infatti, non c'è competitività economica possibile. Occorre trasformare questa battaglia come un fattore di crescita, come un elemento decisivo per mantenere qui i nostri giovani e dare una prospettiva a questo Paese. Invece, la confiniamo nella marginalità come avete fatto voi, perché, pur di fronte alla destinazione di 3,5 miliardi per ridurre il costo del lavoro, non avete messo il Parlamento nelle condizioni di capire come queste misure nel 2024 diverranno strutturali meno. Stiamo discutendo di un DEF che non ha alcun prospettiva nei saldi di finanza pubblica. Partiamo con 12 miliardi in meno solo per evitare che, grazie alle vostre scelte irresponsabili, si aumenti la pressione fiscale sul lavoro. È questa la ragione per la quale non possiamo aprire alcun credito di fiducia nei confronti di questa maggioranza, salvo che non cambi rapidamente strada sui fattori portanti che fin qui l'hanno mantenuta nella propaganda e nel qualunquismo. Quando sento il collega Borghi intervenire - lo dico con grande senso di rispetto, perché tendo sempre ad ascoltare per vedere se un confronto è possibile - trovo che tutta la sua narrazione sia orientata ad individuare un colpevole,

Pensare che sia sufficiente individuare nell'Europa un responsabile per la mancata attuazione delle politiche nazionali un'altra follia, perché tutti sappiamo che oggi abbiamo bisogno di più Europa per affrontare le trasformazioni economiche e sociali. Ci sono alleanze che questa maggioranza dovrà ridefinire per il nostro Paese in Europa, se vuol essere coerente con la parola responsabilità.

e garantire salari maggiori ai nostri giovani, affinché tornino a credere in questo Paese. Guardate che le trasformazioni che abbiamo di fronte sono strutturali.

Lo dico perché, se pensiamo di affrontare il grande tema della denatalità semplicemente annunciando, senza risorse (perché questo è il punto a cui siamo oggi), una riduzione delle tasse una riduzione delle tasse per chi fa figli, stiamo prendendo in giro gli italiani. *(Applausi)*. Stiamo rinviando il problema cercando un colpevole e lo diciamo con tutto l'orgoglio di una forza politica che ha contribuito - perché lì ci sono i nostri valori all'investimento più importante della legislatura precedente, cioè l'assegno unico. Lo diciamo convintamente: guardate che oggi per affrontare il tema della denatalità dobbiamo agire su più fronti e con più ingredienti. la grande questione dell'immigrazione: fino a quando continuerete a considerare l'immigrato un ospite indesiderato, senza diritti, senza affrontare il terreno della cittadinanza, ancora con la stessa impostazione della Bossi-Fini, porterete solo illegalità in questo Paese e non riusciremo a garantire le risorse necessarie per lo sviluppo economico, perché le forze lavoro mancano già tra due-tre anni. Le previsioni dell'Istat ci dicono che il sistema manifatturiero italiano rischia di non avere più le forze lavoro sufficienti per accompagnare la crescita (e parliamo della seconda manifattura europea e tra le prime al mondo in termini di PIL e di occupazione). Bene, a tutto questo voi date una risposta muscolare, negando l'esistenza del problema. Senza un piano straordinario di gestione legale dell'immigrazione, saremo solo costretti a gestire l'illegalità e la criminalità organizzata. Lo dico con grande franchezza, perché qui notiamo anche l'assenza di nuovi servizi per le famiglie e per le donne, che è uno dei punti strutturali. Qui non stiamo dando pagelle al Governo Meloni. Sappiamo perfettamente che sono terreni e nodi strutturali irrisolti da decenni in questo Paese. Quali sono questi nodi strutturali? Abbiamo un basso tasso di occupazione femminile e un alto tasso di disoccupazione giovanile; abbiamo un problema enorme di orientamento e di formazione delle risorse umane, perché la transizione in atto nell'economia e nella società richiede un piano straordinario di formazione permanente; richiede quelle politiche attive delle quali non c'è traccia. Spesso diciamo che sono prerogative e competenze delle Regioni, ma non c'è un'idea del come formare adeguatamente le risorse umane. Senza formazione noi non abbracciamo il futuro. Costruiremo nuova precarietà e nuova solitudine. Aggiungo ancora: di fronte a saldi di finanza pubblica così regressivi, così difficili, come si può ancora vendere l'illusione del "meno tasse per tutti", che spesso è affiancata dal "più evasione per tutti"? Continuo a pensare che dobbiate cambiare strada e aprire un ragionamento serio su una riforma fiscale che è esattamente l'inverso di quello che comunicate ai vostri elettori. A me sorgono dubbi che invece abbiate bisogno di continuare ad alimentare il consenso, accarezzando il pelo all'evasione fiscale, senza garantire invece quel quel diritto fondamentale, quel patto fiscale che lega i nostri cittadini al nostro Paese in base alla quantità di servizi che riusciamo ad erogare. Chi mi ha preceduto ha affrontato molto bene il tema della sanità. Voglio solo fare una considerazione: già oggi abbiamo un problema, ovvero che quel diritto universale alla salute non è più esigibile com'è scritto Dobbiamo fare in fretta a prendere atto che senza una riforma strutturale i cittadini sono costretti a pagarsi le prestazioni sanitarie, perché dopo il Covid - e soprattutto dopo una pandemia questo è ancora più urgente - abbiamo per avere un servizio anche nelle nostre Regioni, a pagarsi una prestazione sanitaria che invece la Costituzione renderebbe universale. Tutto questo richiede un investimento e invece vediamo ritardi sugli investimenti, perché non sapete dove andare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza cercate di far capire che la rigidità dello strumento può metterlo in discussione. Stiamo parlando di mettere in discussione le case della salute, l'unica riforma urgente per tornare a portare nella dimensione territoriale, con i medici di base insieme ai servizi sociali degli enti locali, la protezione indispensabile per evitare che si generi inappropriatezza nei pronto soccorso e nei nostri sistemi ospedalieri. Insomma, state mettendo in discussione gli aspetti fondamentali delle trasformazioni in atto sia nei confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nei confronti di politiche fiscali ed economiche che riteniamo inadeguate. È per questo che non possiamo aprire una linea di credito fino a quando non aprirete un confronto vero sulle riforme, che non sono quell'autonomia differenziata che ci volete far discutere senza oneri per la finanza pubblica, espropriando il Parlamento delle prerogative fondamentali per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per i cittadini. Così non si riducono le aree interne, così si separa l'Italia e si riduce lo spazio per una crescita economica inclusiva, solidale e coerente per garantire un futuro ai nostri giovani.

che nelle Commissioni ognuno di noi dia il meglio di sé e anche in questo caso abbiamo dato il meglio di noi stessi in 5a Commissione per arrivare oggi in Aula. Sono state due ore abbondanti di dibattito in cui sono emersi alcuni spunti particolarmente interessanti a mio avviso, pochi spunti veri fatti con mente e cuore. Sarà che da ventisette anni faccio politica e la faccio sempre mettendoci il cuore e la mente, ma oggi ho avuto difficoltà a

Se siete convinti che in questi sei mesi il Governo Meloni, oltre a essere Mosè, abbia anche ridotto l'Italia in questo modo, c'è qualcosa che non va. Abbiate un minimo di onestà intellettuale, perché, se parliamo di sanità, di scuole e di pubblico impiego, fatevi una domanda, dato che avete governato per decenni. In sei mesi, stiamo cercando di dare una visione alla nostra azione.

quando vi ripresentate alle elezioni negli enti locali, nelle Regioni. Raccontate che quando avete governato per decenni l'Italia non avete consentito al popolo italiano di avere determinate risorse. Raccontate al popolo italiano che non avete avuto visione, perché, se l'aveste avuta, negli ultimi dieci anni, l'immigrazione non sarebbe ai livelli di oggi. Quando il collega Manca, caro Presidente, ci dice che occorre una visione, mi chiedo: la vostra dov'era?

stabilità, credibilità e crescita. Avete raccontato al mondo intero che questo sarebbe stato un Governo non stabile, ma totalmente instabile; e invece vi dimostriamo, giorno dopo giorno, votazione dopo votazione, in Aula e nelle Commissioni, che la maggioranza c'è. Anzi, notiamo che forse qualche problema lo avete voi di minoranza, con passaggi da un partito all'altro (sono capitati anche ieri). Stabilità sociale:

affollano i centri sociali e decidono di contestare il Governo Meloni devastando la propria città. *(Applausi)*. Questa è la stabilità sociale che manca, perché in sei mesi di Governo Meloni - e l'esempio, cari colleghi e caro Presidente, è nei tavoli che portiamo avanti, per esempio, sulle crisi industriali dove noi, come Governo e come maggioranza, ci confrontiamo - spesso è accaduto che sulle crisi industriali che abbiamo ereditato da ministri come Di Maio o altri i sindacati uscissero da quel tavolo con la stessa posizione dell'attuale Governo, e spesso i sindacati non appartengono alla nostra parte politica. Questo piace agli italiani e anche ai mercati, caro Presidente (per suo tramite, lo ricordo al collega Manca). È vero, non dobbiamo rispondere ai mercati: dobbiamo rispondere prima di tutto al popolo italiano, ma i mercati ci danno alcuni indicatori e - a meno

La stabilità economica in questo Documento di economia e finanza è raccontata in maniera chiara, perché cerchiamo una reale stabilità. Non andiamo a raccontare, ma poniamo in essere azioni che hanno una visione politica, una visione politica, che - lo ripeto - è mancata negli ultimi decenni: credibilità. Raccontate di un carrozzone che affossa la nostra Nazione, e invece l'Esecutivo Meloni a testa alta conquista ancora di più gli italiani. Mi piace ribadirlo perché è vero, e voi lo sapete, anche se avete timore di riconoscerlo. Addirittura, si parla di un metodo Meloni, non di un metodo "Giuseppi"

significa parlare d'Italia, di Africa e di Europa con obiettivi che sono l'inclusione, lo sviluppo, la solidarietà e la sostenibilità, cose che noi non abbiamo ereditato da voi, dai Governi Conte I e II, Draghi, Gentiloni Silveri, Renzi e via dicendo.

grave, greve e deleterio e invece il nostro obiettivo e la nostra azione con il DEF sono: il taglio del cuneo fiscale (è poco? Avete ragione, voi non avete fatto manco quello!); la riduzione delle aliquote IRPEF (è poco? Voi non l'avete mai fatta: sono sconti sul costo dell'energia che ancora oggi dobbiamo sostenere, e ci saranno); la crescita demografica (so che a voi non piace questa parola, ma sono azioni sono azioni che voi non avete mai fatto). La crescita demografica è importante non solo ed esclusivamente per la forza lavoro di cui raccontate, per cui grazie agli immigrati potremo avere la sostituzione, ma è importante per tramandare le nostre tradizioni, i nostri sapori e - parlo da sarda - le nostre lingue, i nostri

che ho sentito ieri, se non erro dai 5 Stelle, sul PNRR, secondo cui cerchiamo alibi perché non sappiamo spendere i soldi. No, cari miei, non cerchiamo assolutamente alibi. Lei, Presidente, lo sa, non ha mai cercato alibi facendo politica. Trattiamo i soldi pubblici come fossero i nostri e, quando apriamo una finanziaria, non lo facciamo per pagare una vacanza o comprare un capo firmato.

lo siamo, ma abbiamo degli obiettivi, tra cui quello di essere solidi. Con questo Governo non si raccontano numeri, ma si realizzano obiettivi: fatevene una ragione.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

Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, la sfida finale è quella di gestire un'economia stagnante da circa vent'anni. Qualora riuscisse davvero a portare a meta questi due obiettivi, il suo successo potrebbe essere un modello; a dirlo è Lee Hockstader, in un recente editoriale del «The Washington Post» sul bilancio positivo dei primi sei mesi di Governo del *premier* Giorgia Meloni. Un altro *endorsement* internazionale in risposta ai «profeti di sventura»,

L'analisi del «The Washington Post» prende in considerazione come parametro di successo proprio la politica economica del Governo Meloni, evidenziando l'approccio serio, pragmatico e risoluto con cui è stata scritta innanzitutto la legge di bilancio, cauta per via dell'elevato debito pubblico e volta ad arginare il dramma del caro energia, ma anche altri fatti sorprendenti per l'opposizione, presa in contropiede, ovvero la postura internazionale dopo gli svarioni cinesi del MoVimento 5 Stelle, *ancien régime*, il nuovo ruolo italiano nell'Indo-Pacifico, l'appoggio incondizionato ai valori della NATO e all'Ucraina e la visione strategica del piano Mattei, che il che il Continente africano necessita, passando per una *Faktpolitik* sui migranti, fondamentale soprattutto in un momento storico in cui nell'Unione europea se ne discute finalmente in maniera concreta, con un'*escalation* di sensibilità trasversali. Certamente sarebbe meglio che una parte dell'Europa si rassegnasse all'idea del cambio di *governance* e di politica che i popoli europei stanno attendendo per il prossimo anno ed avesse evitato di zavorrare l'Italia con una sorta di reddito di stabilità, come quello varato ieri dalla Commissione europea. Ma l'Italia della Meloni non strepita e non urla al complotto, anche se l'intervento di certe agenzie di *rating* qualche sospetto lo desta, ma tratta e argomenta in forza della convinzione di un Paese che, nelle difficoltà, ha sempre dimostrato di dare il meglio di sé e di una stabilità di Governo in grado di influenzare le decisioni di Bruxelles, perché il cavallo di razza si vede alla distanza. In questo contesto non possiamo non rilevare come sia più che cruciale il Documento di economia e finanza che discutiamo oggi, che detta la linea del prossimo programma di bilancio e che ancora una volta conferma quella serietà e quella competenza evidenziate dai media internazionali, con cui il Governo Meloni, pur facendo i conti con le annose difficoltà e i vari fronti emergenziali aperti, intende affrontare ancora una volta la programmazione economica. Parliamo di un piano che, sebbene sia ispirato a stime realistiche e prudenti, contiene scelte importanti, che si pongono in linea di continuità con la legge di bilancio che abbiamo approvato qualche mese fa e che ci consente di continuare ad adempiere agli impegni assunti con gli elettori. In breve tempo e nonostante congiunture mai viste in passato, il Governo è riuscito a mettere in campo un'agenda di riforme cruciali per l'ammodernamento del Paese, che rappresentano le fondamenta su cui rilanciare il sistema economico italiano. Il 2023 è una annualità fondamentale per determinare la strada che il Paese intraprenderà nei prossimi decenni. Siamo infatti in un momento di transizione, sia dal punto di vista sociale che politico ed economico. Dobbiamo passare definitivamente da una politica economica di emergenza e di crisi, in particolare quella pandemica e quella della guerra in Ucraina (ma si tratta di una guerra internazionale) ad una politica economica che torni a fare programmazione, capace di implementare iniziative a lungo termine, che sappiano garantire una crescita stabile, solida e duratura, facendo sempre i conti con le variabili che si avvicineranno. Il ministro Giorgetti, nel presentare questo documento, ha sintetizzato perfettamente i capisaldi capisaldi che ispirano l'azione economica del Governo e che emergono indiscutibilmente nel documento che stiamo discutendo: sostegno deciso alla crescita, in modo da poter promuovere il benessere dei cittadini. Non possiamo che condividere le azioni messe in campo, dai nuovi interventi in favore delle famiglie, in particolare per quelle numerose, a quelli in favore delle imprese, alle misure destinate a rilanciare gli investimenti e rafforzare la competitività del Paese. Va peraltro evidenziato come il Governo, nella fissazione e nell'attuazione degli obiettivi, abbia mantenuto alta l'attenzione sulla sostenibilità dei conti pubblici, impegnandosi anche ad una graduale riduzione di *deficit* e debito, in previsione anche della riforma del Patto di stabilità e crescita, puntualmente varata ieri dalla Commissione europea, che ci consente flessibilità, ma ci richiede nuovo rigore nel rientro sul debito. Questa è serietà, questo è perseguire l'interesse nazionale. Sono orgogliosa di far parte di questa maggioranza, che si dimostra responsabile, rispettando gli impegni assunti, senza scaricarne gli oneri sulle future generazioni. Questa affidabilità, nonostante gli auspici contrari delle parti più radicalizzate dell'opposizione, è stata riconosciuta, come abbiamo detto, a livello internazionale, sia dal mondo politico che da quello economico. Si badi bene: essere responsabili non significa non essere coraggiosi e questo lo si è dimostrato in un momento come quello attuale, in cui domina l'incertezza, non solo attraverso gli oltre 4 miliardi di euro messi in campo per le misure espansive, ma soprattutto attraverso le ulteriori risorse che sono state destinate alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori a reddito medio-basso. Dopo anni di oppressione fiscale questo Governo segna la discontinuità e, invece che mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ha il coraggio di impiegare le maggiori risorse in via prioritaria nel taglio della tassazione, nonostante l'Unione europea tenda a non aiutarci. Sono apprezzabili anche le misure a favore delle imprese, che abbiamo discusso in 9a Commissione e che riguardano in particolare la proroga proroga per il 2023 del credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Mezzogiorno, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, le risorse stanziate per importanti progetti di comune interesse europeo e l'incremento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Presidente, Ministri, i segnali ci sono e sono positivi. In questi anni il sistema economico italiano si è dimostrato resiliente, rispondendo bene alle situazioni contingenti e reagendo meglio di molti nostri *partner* europei con molto meno debito pubblico. L'aumento delle previsioni di crescita per l'anno in corso è il nostro primo importante risultato e ci consente di poter agire con più forza e autorevolezza anche a livello comunitario. Questo nuovo clima di fiducia è attestato anche dalla significativa ripresa dei consumi delle famiglie. L'industria manifatturiera e quella industriale hanno dato segnali di espansione, il settore delle costruzioni, dell'auto, dei servizi e della cultura sono ancora in crescita. La ripresa La ripresa del turismo sta contribuendo a rilanciare il comparto del commercio e il settore alberghiero e ristorativo, che è tornato al di sopra dei valori pre-crisi. Sta a noi ora saper valorizzare questo clima positivo, riscontrando la fiducia dei mercati e degli italiani. Dovremo cogliere tutte le opportunità che questo periodo ha portato con sé, in particolare proseguendo nella realizzazione di di tutte le misure previste dal PNRR, come ha detto ieri il ministro Fitto, che è un punto fondamentale non solo per l'ottenimento dei fondi, ma anche e soprattutto per la realizzazione delle riforme strutturali che da tempo il Paese aspetta per volare. Certo - come diceva il premio Nobel Modigliani, ripreso dal ministro Giorgetti - dal conteggio del debito si sarebbero dovuti escludere ieri, nella Commissione europea, gli investimenti del PNRR, inserendo quella che in gergo viene chiamata *golden rule*, ovvero la possibilità di contabilizzare in modo diverso, ai fini della sorveglianza di bilancio, gli investimenti che uno Stato fa in determinati settori. Ma supereremo anche questo. Abbiamo ancora qualche mese per lavorare sulla prossima legge di bilancio e io voglio esprimere un auspicio, ovvero che si superi questo clima di divisione e balcanizzazione politica. Dobbiamo lavorare insieme, nel rispetto nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, ma contribuendo tutti a dare insieme le risposte che gli italiani si aspettano, perché per rilanciare il sistema Paese in modo duraturo sono fondamentali la coesione politica e la collaborazione più ampia possibile tra le istituzioni. Noi ci siamo e siamo pronti a farci promotori di un dialogo costruttivo e positivo, a condizione che si abbandonino la *bagarre* e gli attacchi strumentali finalizzati alla crescita di un punto nei sondaggi, che non danno alcun valore aggiunto al dibattito politico. Ad ogni modo, anche se vi dovesse essere l'indisponibilità da parte delle opposizioni a questo percorso, ci tengo a rassicurare gli italiani. Questo Governo andrà comunque avanti con la stessa forza, decisione e convinzione che lo lo hanno contraddistinto e che derivano dalla legittimazione che gli elettori continuano ad accordargli in tutte le tornate elettorali. Forse la cattiva notizia - prendo sempre in prestito le parole del «The Washington Post» - per certa opposizione è che sarà difficile duplicare la sala segreta di acume, buon tempismo e fortuna del *premier* Meloni e

e finanza - a nostro avviso - deve essere la cartina di tornasole del messaggio che si dà al Paese. Stamattina chiudevo il mio intervento dicendo che il punto principale la coesione sociale e la riduzione delle disuguaglianze e come affrontare questo tema. In questo DEF tutto tutto questo non c'è e manca una visione. Sento molto spesso, dai colleghi della maggioranza, dire che il Governo durerà. È un Governo politico e io ho rivendicato altre volte che sono molto contento che una volta tanto ci sia un Governo politico, perché si deve assumere le sue responsabilità.

già previsto dal Governo precedente (quindi si arriva a 10 miliardi). In questo Documento non si dice, ma il prossimo anno bisogna trovare 12 miliardi per mantenere lo stato attuale.

le imprese. Occorre costruire un meccanismo che sia in grado di recuperare il potere d'acquisto di salari e stipendi.

in molte famiglie del Nord, in questo caso, lavorano le badanti, magari in nero, che non si mettono a libro paga e sono senza diritti.

parliamo di favorire l'occupazione, quella buona. Cosa c'è sulla questione della riduzione della precarietà? Vi sfido a leggere il DEF, leggiamolo tutti insieme: non c'è una virgola sulla riduzione della precarietà. Questo è il dato fondamentale. Se noi vogliamo mantenere i nostri giovani, dobbiamo dare loro un giusto salario, mentre oggi sono sottopagati, una prospettiva nel lavoro che fanno, soprattutto

perché dobbiamo tendere a una società che sia più coesa e più sicura, perché solo così diamo sicurezza. con la coercizione, ma con la partecipazione e con il coinvolgimento: questo è il dato su cui dobbiamo investire per il futuro. Per questa ragione, credo che sia un fatto estremamente positivo che in questo caso

il quadro delineato dal DEF è stato definito prudente, equilibrato e condivisibile, per quanto riguarda sia il quadro macroeconomico, sia quello di finanza pubblica.

Le previsioni su cui poggia il DEF possono essere smentite anche repentinamente dall'aggravarsi dei vari fronti geopolitici come un'*escalation* dell'aggressione russa all'Ucraina, il permanere dell'inflazione di fondo su livelli elevati, l'irrigidimento delle condizioni di finanziamento dei principali Paesi avanzati e, non ultimi, i recenti episodi di dissesto bancario. Esistono, inoltre, fronti di rischio specifici nei contesti europeo e nazionale, come il prezzo dei prodotti energetici. È pur vero che il prezzo del gas è sceso da una media annua di 235 euro a una di 45 euro megawatt/ora, ma rimane pur sempre al di sopra del livello dei prezzi pre-crisi energetica. Inoltre, il taglio della produzione di petrolio deliberato dall'OPEC indica come prudente il non considerare terminata la fase di volatilità dei prezzi dei prodotti energetici. Allo stesso tempo, anche le politiche monetarie della BCE per contrastare l'inflazione potrebbero incidere ulteriormente al rialzo sui tassi di interesse. Sul fronte della finanza pubblica va considerato che a fine 2023 sarà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita. È quindi importante che gli Stati membri recepiscano sin d'ora alcuni dei principi della proposta di riforma della Commissione UE come l'obbligo di garantire che il rapporto tra debito pubblico e PIL sia in discesa verso l'obiettivo di medio termine, oppure garantire il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL nel medio termine. Alla luce di ciò, i pur prudenti andamenti degli indicatori dell'orizzonte 2023-2026 e il confronto con gli andamenti tendenziale e programmatico e anche il confronto tra gli andamenti programmatico NADEF con programmatico DEF non lasciano grandi spazi di manovra. Infatti, nonostante il quadro macroeconomico più favorevole delle attese, i saldi di finanza pubblica a legislazione vigente sono solo leggermente migliori rispetto ai programmi dello scorso anno. In particolare, l'indebitamento netto e il rapporto debito-PIL vanno tenuti sotto stretta osservazione. Con riferimento all'indebitamento netto, è necessario ricordare il nuovo trattamento statistico dei crediti di imposta edilizi che passa dal criterio di competenza a quello di cassa; un cambio di criterio che modifica il profilo temporale dell'indebitamento netto, ma che non muta la sostanza di un disavanzo accresciuto del triennio di oltre 90 miliardi. Fatta questa premessa, l'andamento dell'indebitamento netto nell'orizzonte di previsione presenta valori pressoché uguali tra NADEF, DEF tendenziale e DEF programmatico e la graduale riduzione verso l'obiettivo del 3 per cento che si prevede verrà raggiunto nel 2025. Il Governo sceglie inoltre di non utilizzare il lieve miglioramento dello 0,15 per cento, pari a circa tre miliardi, per ridurre l'indebitamento netto. Sceglie invece di destinarlo invece a una riduzione temporale dei contributi sociali a carico dei lavoratori con reddito medio-basso; un intervento temporaneo, tanto che a partire dal 2024, per evitare un aumento della pressione fiscale, dovranno essere reperite ulteriori risorse che peraltro, ad oggi, non si leggono nel DEF. Queste serviranno per rendere strutturali o almeno per prorogare sia tale nuovo intervento sui contributi sociali, sia gli interventi già in essere e previsti nella legge di bilancio per il 2023. Il DEF peraltro stima che gli oneri connessi alle politiche invariate ammontino allo 0,3 per cento del PIL nel 2023 per oltre 9 miliardi e allo 0,4 per cento del PIL nel 2026 per oltre 12 miliardi. non lascia intendere chiaramente dove verranno reperite le nuove risorse, limitandosi a un generico richiamo al rafforzamento della revisione della spesa pubblica e a una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente, dimenticando in quest'ultimo caso che il fondo per il recupero dell'evasione dovrebbe essere destinato a finanziare la riforma fiscale e non genericamente a rifinanziare le politiche invariate. È altresì evidente che il DEF non individua gli spazi per finanziare alcuna delle promesse elettorali del Governo né sulla riforma fiscale né sul superamento lo reputo insostenibile - della legge Fornero, ma nemmeno per gli urgentissimi interventi sul *welfare* e sulla sanità. Anzi, sotto questo profilo, gli analisti confermano che la spesa sanitaria

una prospettiva incompatibile con le necessità del Sistema sanitario. Condivido pertanto la preoccupazione: prima di ogni eventuale aumento di spesa o riduzione di entrata rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, devono essere identificate le coperture adeguate strutturali e credibili. Tra queste, un impegno dovrebbe essere rivolto al ripristino di Opzione donna, con i requisiti in vigore nel 2022, e quindi un'anzianità di almeno trentacinque anni di contribuzione e di almeno cinquantotto anni di età, cinquantanove per le autonome. tenere conto che lo strumento di Opzione donna, trattandosi di pensione contributiva, è interamente a carico di chi ha versato i contributi, ricevendo di fatto chi opta per Opzione donna - i contributi sulla base di un calcolo completamente contributivo, che porta ad ottenere in base a quello che si è realmente versato. versato. L'intervento su Opzione donna porterebbe un forte contributo al riassorbimento delle differenze di genere, come vuole il PNRR, in questo caso dando una risposta alle alle differenze retributive e contributive che da anni colpiscono la vita lavorativa delle donne, o meglio di una sola donna su due che in Italia lavora. Con riferimento al rapporto debito pubblico/PIL, il DEF conferma una riduzione, seppur lenta: nel 2026, al termine dell'orizzonte di programmazione, il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere al 140,4 Il calo complessivo di quattro punti rispetto al 2022 dipende da un differenziale favorevole tra la crescita nominale del prodotto, l'onere medio del debito e la persistenza di un avanzo primario superiore al 2 La riduzione del rapporto debito/PIL non è, però, automatica in assenza di precisi interventi. Per prima cosa, l'onere sul debito è destinato ad alzarsi perché l'aumento dei tassi di interesse, già deciso dalla BCE e probabilmente in ulteriore rialzo, è mitigato per ora solo dalla vita media residua del debito pubblico italiano relativamente alta e pari a circa sette anni. Tuttavia, secondo le simulazioni presentate nel DEF, anche se gli obiettivi fissati venissero pienamente raggiunti, in assenza di un'ulteriore correzione dei conti, il rapporto tra debito e PIL tornerebbe ad aumentare già negli anni immediatamente successivi al 2026. È di tutta evidenza che, per evitare tale insostenibile scenario, le politiche di bilancio dovranno mantenere adeguati avanzi primari e spingere una crescita economica con tassi di crescita vicini all'uno obiettivi non raggiungibili senza una precisa determinazione a risolvere alla radice due principali ostacoli: in primo luogo, il recupero di efficienza ed efficacia del sistema Italia, che garantisca la produttività dei fattori, lavoro e capitale, con il superamento delle storiche criticità criticità e quindi la messa a terra di tutte le riforme previste, dalla giustizia alla pubblica amministrazione, dal fisco alle politiche attive del lavoro, alla digitalizzazione; in secondo luogo, l'inversione di tendenza del calo demografico, da compensare nel breve termine con l'immigrazione e nel medio termine con la natalità. La natalità è diretta conseguenza del protagonismo femminile, come confermano tutti i dati dei Paesi europei più performanti. Per concludere, signor Presidente, questo DEF non lascia scampo a una rotta laboriosa e determinata, quella per la messa a terra di tutti gli interventi, gli investimenti e le riforme del PNRR. Solo così riusciremo nell'obiettivo della modernizzazione del Paese e del superamento dei ritardi strutturali e delle diseguaglianze generazionali, territoriali e di genere e per lasciare alle prossime generazioni un Paese più giusto e un tessuto più economico più competitivo. Per questo, come Gruppo Per le Autonomie esprimeremo un voto favorevole per le risoluzioni che indicheranno in modo inequivocabile il raggiungimento di questi obiettivi. Signor Presidente, io penso che sia giusto inquadrare la discussione del DEF in uno scenario geopolitico, che è davvero comprensibilmente ed obiettivamente complesso. tempi di guerra, scatenati dalla Russia con l'invasione dell'Ucraina, sono sicuramente aumentati. C'è una tensione in Oriente nel rapporto tra Cina e Taiwan; c'è un recupero, da parte della Cina, di un ruolo di dimensione globale, in netto contrasto con l'Occidente, per una evidente competizione di supremazia mondiale. E c'è anche, dal punto di vista economico, una ripresa, dopo il Covid-19, del ruolo della Cina. Il quadro è, quindi, complesso. Nessuno di noi vuole fare finta di non comprendere appieno le dimensioni e la portata delle difficoltà che ci sono. È vero anche che ci sono dei cambiamenti, che vanno compresi e monitorati fino a fondo. Penso, per esempio, al tema della logistica mondiale. Noi abbiamo un cambiamento, se vogliamo anche epocale e di indirizzo, da una dinamica orizzontale ad una dinamica verticale, che non possiamo sottovalutare. Abbiamo anche avuto un miglioramento, di cui dobbiamo dare atto a chi ha governato prima di questo Governo, cioè Mario Draghi, dei flussi di gas tra la Russia e l'Europa, che sono stati progressivamente sostituiti col Medio Oriente e con il Nord Africa. Bisogna conoscere che cosa sta succedendo nel mondo. C'è una

quindi, che per diverse ragioni (gas, logistica, rotte) può riconfigurare un ruolo importante e centrale del Mediterraneo e può rilanciare il ruolo che, che, per nostra natura, è tipico, insito nel sistema italiano, della piattaforma logistica del nostro Paese. Parto da qui perché una delle questioni su cui penso che dovremmo cercare di capire meglio la strategia del Governo è il tema del tanto tanto sbandierato Piano Mattei: un nome suggestivo, un nome che ci piace, ma vorremmo anche capire quali sono le azioni reali che il Governo sta intraprendendo per metterlo in atto.

alle persone incaricate all'interno delle società, tra cui sicuramente l'ingegner De Scalzi, che anche voi evidentemente apprezzate per il lavoro svolto. Questo Piano, però, rimane un'araba fenice: che vi sia ciascun lo dice, ma dove sia nessun lo sa. E non serve scomodare Mozart per capire che siamo in presenza di un enigma, un enigma che, che, ormai, meriterebbe di essere compreso. *(Applausi)*. Insomma questo è un Governo che capisce poco i processi mondiali, se ne occupa molto poco, anche perché isola costantemente il nostro Paese in ambito europeo. Tuttavia, se può, fa continuo ricorso alla retorica degli scenari apocalittici, anche per esempio sul tema della crisi demografica, anche per esempio sul tema della crisi demografica, anche quando questo riguarda la richiesta urgente di domanda di lavoro delle imprese. Se, però, con la mano destra fa questo, con la mano sinistra

Guardiamo allora ai dati veri di questo Documento, che ha innanzitutto un'incapacità di risoluzione del problema del debito, del debito, che rimane una zavorra per il nostro Paese: non parlo - come dice sempre la collega Fregolent, citando il nostro ex presidente Mario Draghi - del debito buono, ma del debito che non genera investimento e crescita. Questo DEF Questo DEF configura la spesa sanitaria sotto il 7 per cento del PIL e quindi un'emergenza reale e forte del Paese non è risolta all'interno di questo Documento. C'è una sottovalutazione dell'impennata dell'inflazione, del costo delle materie prime, dell'aumento del costo del denaro, della diminuzione degli investimenti, del costo dei mutui. In sostanza, quella che si va profilando è una crescita bassissima, che non produce né il risultato di una riduzione reale del debito, né una capacità seria di investimenti e di ridistribuzione. *(Applausi)*. È la matematica a dirlo, oltre che la logica. allora che non si possa non parlare di un DEF inadeguato e che sia anche nostro dovere farlo. Noi siamo un'opposizione che fa proposte, che vi sfida sulle questioni, che anche sul PNRR ha avuto un atteggiamento costruttivo.

del tema della diminuzione delle accise. Non c'è traccia della riforma delle pensioni - vi terrete la Fornero a lungo, nonostante i proclami televisivi - e non non c'è traccia di una riforma adeguata di politica fiscale. Non c'è traccia neppure di una strategia sulla sofferenza demografica. Nell'ultimo anno sono nati 400.000 bambini C'è un aumento dell'età media e le conseguenze sono evidenti. Il rischio è il collasso del sistema pensionistico, del sistema produttivo, del sistema sanitario e del sistema formativo. Si può anche continuare a fare propaganda, ma, siccome all'epoca di Draghi la crescita in questo Paese c'è stata, la propaganda è a zero. È a zero, se non ci sono iniziative, se non c'è una capacità di mettere in campo una visione comprensibile sulle politiche migratorie, sulle politiche dei flussi, sulle politiche del lavoro e fiscali, sulle politiche della giustizia, su cui ancora non si è capito dove volete andare a parare, e sulle politiche demografiche.

la discussione che abbiamo fatto ieri, e cioè la discussione di una maggioranza che dice in maniera chiara e cristallina che non è in grado, non è capace di spendere le risorse del PNRR *(Applausi)* e che non lo è non perché il lavoro consegnato è insoddisfacente. Non è in grado perché in questi sei mesi non ha saputo mettere in campo un sistema di semplificazione e velocizzazione delle opere; non ha saputo riformare la pubblica amministrazione; non ha saputo aiutare i Comuni e cambiare i progetti che erano in grado di partire. Con questo non voglio dire che tutto fosse meravigliosamente a posto; certo, c'erano delle criticità, ma non si capisce come mai voi queste criticità, anziché affrontarle il primo giorno di insediamento di questo Governo, le avete prese in mano dopo sei mesi. Per quale motivo, a fronte della possibilità di dare una svolta, c'è qualche Ministro, per esempio il ministro Salvini, che continua a ricordare che tutto sommato quelle risorse possono anche non essere spese? Voglio rammentare a tutti voi che non spendere quelle risorse, dimostrare l'incapacità di visione, ma anche operativa del nostro Paese, è una grande sconfitta, una grande resa per l'Italia *(Applausi)*, un colpo duro a una visione europea più solidaristica che noi dobbiamo auspicare vada avanti, non che torni indietro. Cosa proponiamo? Noi innanzitutto vi chiediamo di guardare un po' indietro rispetto agli anni in cui questo Paese cresceva. Il Governo Renzi potrebbe essere un buon esempio per voi. Potrebbe ricordarvi, per esempio, che con Industria 4.0 e con Italia sicura, noi abbiamo fatto delle cose importanti: investimenti in macchinari, impianti, mezzi di trasporto, digitalizzazioni, gli interventi strutturali che consegnano al Paese un vantaggio competitivo, mettendolo nella condizione di essere davvero moderno in Europa e nel mondo. Sul tema delle politiche

più convincenti rispetto a quello che avete provato a fare. In sostanza è chiaro che il nostro profilo come opposizione - parlo di Azione-Italia Viva - continua a essere quello di forze politiche che che tifano sempre per il Paese, che cercano di dare una mano in termini di proposte, che sono convinte che il Paese possa farcela, ma che non possono esimersi da una critica dura molto severa rispetto a questi mesi di Governo. E questa critica severa si tradurrà - io credo in maniera molto coerente - da un lato, con l'assunzione di responsabilità piena nel voto sullo scostamento, augurandoci tutti quanti che non serva solo a generare debito, ma serva anche realisticamente a dare una mano a politiche operative; dall'altro lato, però, con un voto pienamente e convintamente negativo sulla risoluzione della maggioranza che in qualche modo riassume e riepiloga lo strumento del DEF che - come abbiamo detto - reputiamo inadeguato, reputiamo inadeguato, ma soprattutto senza alcuna visione strategica.

quello che ci accingiamo a votare oggi in Assemblea è il primo Documento di economia e finanza interamente frutto delle scelte di politica economica del Governo Meloni e della maggioranza di centrodestra. È utile anche ricordare, visto che abbiamo ascoltato in quest'Aula tanti

con grande coraggio e con scelte che abbiamo già identificato nella manovra precedente, abbiamo tracciato una linea e una

però ormai un paio di anni che lo facciamo: per 8 miliardi di euro nel 2021, lo scorso anno, nella manovra finanziaria, abbiamo tagliato di 3 punti il cuneo fiscale e oggi lo facciamo con altri 3,5 miliardi di euro. Questi sono dati importanti, che testimoniano l'impegno che la maggioranza e il Governo stanno mettendo oggi a punto, per sostenere i lavoratori e non solo, ma anche e soprattutto le imprese, per liberare risorse che servono oggi alle imprese, per creare lavoro. Nel 2024 abbiamo anche a disposizione, come è scritto nel DEF, 4,5 miliardi di euro, che servono per un altro caposaldo di questa maggioranza, ovvero la riforma fiscale, che il Governo ha subito messo in campo nei primi mesi della legislatura e che ha già iniziato il suo *iter* e il suo percorso legislativo nelle Aule parlamentari. Si tratta di un altro impegno forte del Governo. È importante ancora evidenziare che è prevista la riduzione della pressione fiscale, da sempre un cavallo di battaglia di Forza Italia e del centrodestra: dal 43,3 per cento nel 2023, prevediamo una decrescita appunto della pressione fiscale, con una riduzione al 42,7, nel 2026, e lo stesso vale per il debito, che scenderà di altri 4

della nuova politica economica del Governo. Il Governo si trova a varare oggi un Documento di economia e finanza

che abbiamo oggi di fronte a noi e per ricordare quale è oggi l'incertezza del futuro, perché non ci sono, anche da un punto di vista economico, dei punti di riferimento. Occorre evidenziare che la guerra e il Covid hanno portato ad una crescita importante dell'inflazione.

quindi si articola e si delinea su tre principi fondamentali e su tre obiettivi che definisco programmatici.

si eliminano tutte queste misure, ma si continuano a individuare delle misure permanenti di sostegno alle famiglie e ai soggetti più vulnerabili. In secondo luogo, abbiamo la riduzione graduale del *deficit* e del debito della pubblica amministrazione rispetto al prodotto interno lordo. c'è il sostegno alla ripresa dell'economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere degli italiani che siano più elevati rispetto al decennio passato.

con la riduzione e il taglio delle spese dei Ministeri: un miliardo e mezzo nel 2023 e due miliardi nel 2025. Il quadro degli strumenti per la crescita non si ferma qui. Ne abbiamo parlato tanto in queste settimane in quest'Aula, anche ieri: l'utilizzo di tutti i fondi del PNRR che farà non soltanto crescere il prodotto interno lordo, ma ridurrà il tasso di disoccupazione nel nostro Paese in questi anni. Questi sono fatti concreti con i quali l'opposizione si deve confrontare. Molto importante è anche, e non per ultimo - Presidente, mi dia solo un minuto per concludere - il quadro delle riforme che abbiamo messo in campo, con la principale di esse, la riforma delle riforme, quella fiscale, che ha già iniziato il suo *iter* parlamentare. Con questo vi dovete confrontare. Forza Italia ha già espresso il suo voto in Consiglio dei ministri, votando favorevolmente, perché la strada intrapresa dal Governo getta le basi per la manovra finanziaria che andremo a fare nel prossimo dicembre 2023, 2023, in sintonia soprattutto con gli obiettivi del nostro programma, che - lo voglio ricordare - è stato votato dalla maggioranza degli italiani.

per il nostro Paese. *(Applausi)*. Ecco perché solo con questi strumenti riusciamo a combattere la crisi economica che, ahimè, in questi anni ci ha distrutto e messo in grande difficoltà. È per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il Documento di economia e finanza in discussione, il primo - come è stato ricordato - a firma del presidente Meloni e del ministro Giorgetti, dimostra tutta la pochezza e l'incapacità dell'attuale Governo *(Applausi)* di dare risposte alle diverse emergenze e priorità del Paese. Con meri espedienti lessicali, l'Esecutivo e il Ministro dell'economia e ambizioni responsabili, prudenza fiscale e pragmatismo, nel tentativo di nascondere il prosaico significato di questi termini, ovvero: austerità e tagli. In più, con un'operazione ardita, illogica ed economicamente folle, nelle premesse al DEF si pone come obiettivo - peraltro annunciando e definendo un principio economico nuovo che il Governo ha coniato - la moderazione salariale, che secondo il Governo dovrebbe servire a contrastare il pericolo di una spirale prezzi-salari. Il tutto quando i più autorevoli osservatori, a partire da alcuni banchieri centrali della BCE come Fabio Panetta e Isabel Schnabel,

proprio nei giorni scorsi Eurostat ha certificato che nel 2022 l'Italia è il penultimo Paese in Europa quanto al recupero dell'inflazione.

in Italia l'incremento è stato appena del 2,3 per cento. Questo senza considerare che in Italia i salari sono fermi da oltre vent'anni e l'OCSE ci dice che c'è stata una perdita per cento. Di fronte a questa emergenza, sia economica che sociale, il Governo Meloni cosa fa? Parla di moderazione salariale. Ci chiediamo: ma dove vive l'Esecutivo? Si è scelta una politica economica di rigore e marcatamente restrittiva. si programma un draconiano abbattimento del rapporto *deficit*-PIL in calo dal 5,6 per cento del 2022, al netto delle riclassificazioni contabili, al 2,5 per cento si punta su una crescita economica che noi abbiamo definito da prefisso telefonico, prevista dal Governo all'1 per cento

difficilmente conseguibile con un *trend* di crescita così modesto, tranne se non si ricorre, come avete deciso di fare, ai tagli alla spesa.

3,4 miliardi, appena lo 0,15 per cento del PIL, dato dalla differenza tra *deficit* tendenziale 2023 (4,35 per cento in rapporto al PIL) e *deficit* programmatico, confermato al 4,5 un mini margine fiscale che si ha avuto il coraggio di spacciare per tesoretto, ma che potrebbe semplicemente derivare dal recente cambiamento contabile di Eurostat. Questi sono, in sintesi, i numeri di una manovra che il Governo ha definito, in alcune uscite pubbliche e interventi sulla stampa, "espansiva"; lo avete anche riferito qui in Aula quando invece i dati dimostrano in maniera inequivocabile tutt'altro. Dimostrate anche di non conoscere i dati della manovra, perché quando il presidente Meloni afferma, com'è accaduto in una recente intervista su «Milano Finanza», di voler ridurre il debito pubblico con la crescita economica, sconfessa se stessa, viste le prospettive economiche così desolanti e misere. La verità è che il Governo Meloni ha sposato e ha anticipato forse la politica dell'*austerity*, fatta di tagli alla spesa e di scarsa prospettiva economica, così come comprovato dal ritorno all'avanzo primario, per cento del 2022 passerà a + 2 per cento entro il 2026. Questo significa realizzare una stretta fiscale fatta di tagli alla spesa corrente e soprattutto - ahimè - agli investimenti stimabile in oltre 60 miliardi a valori attuali: altro che ridurre il debito pubblico con la crescita economica. Questi sono numeri da vacche molto grasse; anzi, per noi magre, per voi grasse. È una stretta di cinghia che difficilmente il Paese potrà sostenere sul piano sociale ed economico, in considerazione anche della manovra correttiva di 15 miliardi che Bruxelles ha già comunicato con la nuova letterina che è arrivata a seguito della riforma del Patto di stabilità, proprio in base a quello che voi avete certificato nel DEF. Qui si rischia, caro Governo, di entrare nuovamente nella trappola del debito, già sperimentata a partire dall'ultimo Governo di centrodestra del 2009 e che gli italiani ricordano ancora. Questa descritta è la verità inconfutabile dei numeri che questo Governo ometterà sempre di dire ed ammettere, preferendo ancora una volta la sola propaganda. L'approvazione di questo DEF 2023, inoltre, segna la definitiva rottura con le aspettative di crescita economica del Paese e fa calare un triste sipario sulle politiche espansive del Governo Conte 2, che hanno permesso al rapporto debito-PIL di ridursi di ben 13 punti e alla crescita economica del PIL di raggiungere la cifra *record d*i quasi l'11 Entrando nel merito del DEF, avete deciso di nascondere, come polvere sotto il tappeto, i veri problemi dei cittadini e delle imprese. Ne cito solo qualcuno per motivi di tempo, a titolo esemplificativo: ad esempio, l'impoverimento delle famiglie e l'emergenza salariale. Soprattutto su questi aspetti avete annunciato un misero taglio al cuneo fiscale di 3,4 miliardi, che corrispondono a pochi spiccioli di 9 e 16 euro, peraltro solo per il periodo di maggio-dicembre. una misura che riteniamo insufficiente, perché in Italia non c'è solo il problema di tagliare le tasse sul lavoro, ma è necessario aumentare i salari poveri, introducendo il salario minimo legale *(Applausi)*, adeguare gli stipendi all'inflazione, così come stanno facendo Germania, Francia e Spagna. Cosa aspettate a farlo? Questo aiuterebbe anche molti settori nella ricerca dell'occupazione, favorirebbe la natalità e soprattutto eviterebbe il rischio prossimo del crollo dei consumi, del mancato pagamento dei mutui e della sfiducia delle imprese. Sulla natalità, caro Ministro, attendiamo di conoscere la proposta che ha annunciato. In base ai nostri calcoli, costerà 80 miliardi, ma attendiamo adesso di sapere effettivamente qual è la proposta. Sulla sanità pubblica fate un taglio di risorse rispetto al PIL che passeranno dal 7 per cento al 6,7 per cento, una situazione inaccettabile che metterà a rischio il diritto universale alla salute. Si tagliano le pensioni di 10 miliardi, rimandate la delega fiscale e rimandate il superamento della legge Fornero, due cavalli di battaglia che avete promesso di portare costi quel che costi (queste erano le parole di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini). Ancora una volta i numeri reali smentiscono i vostri conti, ma mi chiedo: dov'è il buco di bilancio che avete più volte ribadito? Nel DEF c'è scritto che il fabbisogno di cassa addirittura si è ridotto di 40 miliardi. Ma vi rendete conto di quante fesserie sono state dette sul superbonus e sugli effetti del superbonus? *(Applausi)*.

sono come sabbie mobili che, viste da lontano, sembrano solide e sicure, ma si rivelano inconsistenti e insidiose da vicino». Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla proposta di risoluzione della maggioranza sul DEF, in considerazione delle tematiche che vi vengono

Dite che rimandate tutto a degli spazi fiscali: 4 miliardi avremo per il 2024. Proseguite poi sul tema del lavoro, che limitate al solo cuneo fiscale, ma - attenzione non c'è solo il problema del cuneo fiscale, c'è il problema di ridurre il costo del lavoro per le imprese e di indicizzare i salari. Parlate di occupazione, ma quale occupazione? Noi vogliamo un'occupazione di qualità, quindi no alla precarietà e soprattutto salari dignitosi, perché senza questi non riusciamo a risolvere l'altro problema a voi caro, che è quello della denatalità. Senza la stabilità del lavoro e senza redditi dignitosi, il tema della natalità non lo si può risolvere solo con qualche mancia o con qualche sussidio.

il Documento di economia e finanza che andiamo ad approvare è in linea con la legge di bilancio approvata dal Governo Meloni di centrodestra che, come questo documento, era una manovra molto semplice, solida, pragmatica, seria, esattamente quello che va fatto in un momento di particolare incertezza come quello attuale. Non nascondiamoci dietro a un dito: i costi dell'energia, i tassi di interesse, la modifica del Patto di stabilità europeo sono tutti elementi che vanno considerati con la massima attenzione. Ricordiamo le polemiche infinite sulla legge di bilancio: non c'è abbastanza per i costi dell'energia, e invece i fatti ci hanno dato ragione ed è stato fatto quello che andava fatto, sono state concentrate in un periodo perché poi bisognava vedere l'evolversi della situazione, altrimenti si sarebbero buttate via risorse. Ricordiamo i fiumi d'inchiostro per la fine dello sconto statale sui carburanti: anche in quel caso sembrava che venisse giù il mondo, e invece si è evitato di buttare via fiumi di risorse pubbliche, perché poi i costi sono rientrati da soli. Ecco, questo è quello che va fatto in un momento particolarmente incerto e complesso come questo: proseguire, passo dopo passo, su basi solide, quindi aggiornando di volta in volta le politiche economiche sulla base dei dati che si aggiornano in tempo reale. Intanto, tra l'altro, l'Italia cresce più del previsto. Sappiamo tutti che il Documento di economia e finanza non è la Bibbia con cui si scriverà la legge di bilancio. È evidentemente frutto di una stagione di incertezza; il vero documento sarà la NADEF, la Nota di aggiornamento al DEF dopo l'estate, e lì ci saranno i dati giusti per poter fare la prima legge di bilancio di legislatura del Governo di centrodestra. Questo è il punto. Questo è un documento ponte, che programma a medio termine, sì, ma il documento vero sarà quello di Nel frattempo, cosa fanno Governo e maggioranza? Stanno fermi? No, perché nel mentre ci sono anche riforme che creano PIL, creano sviluppo e non necessariamente hanno bisogno di risorse e di stanziamenti. Tra l'altro, tutte le risorse disponibili sono state giustamente assegnate alla priorità delle priorità, che è il costo del lavoro per i redditi più bassi. Ora, che vi lamentiate anche di questo è onestamente paradossale!

il magazzino fiscale, cioè, imposte e tasse che lo Stato non riesce a incassare. Erano 810 miliardi a fine 2018,

Ma se una partita IVA, se un contribuente fa ricorso, e una volta su due vince lui e perde l'Agenzia delle entrate, vuol dire che c'è un problema, che non funziona neanche l'accertamento.

Questo per i fatturati più bassi. Poi, per i fatturati medio bassi e medio alti, per la fascia intermedia, il concordato preventivo biennale. Oggi l'Agenzia delle entrate ha tutti i dati puntuali per arrivare a capire, azienda per azienda, qual è il giusto fatturato. C'è tutto: c'è la fatturazione elettronica ed abbiamo tutti i dati. Si dice che cosa si vuole fatturare. Fatturi di più? Buon per te. Fatturi di meno? Peggio per te. Però, regole semplici e non più lo Stato di polizia che dà dell'evasore a prescindere a chi sbaglia, magari facendo errori formali. Poi, per le aziende più grandi, è previsto il *corporate compliance.*

Allora va rivisto il mercato del lavoro. Anche in questo caso, il 1° maggio il Governo varerà un decreto che rimuoverà un po' di ostacoli. Poi vi è la questione del reddito di cittadinanza. Se funzionava così bene, come mai non c'è incontro tra domanda e offerta di lavoro? lavoro? Oggi l'INPS ci dice che nel primo trimestre ci sono state 300.000 domande, con un calo, su base annua, del 25 per cento, solo mettendo qualche paletto. Queste sono tutte risorse in meno che lo Stato spende e che possono essere giustamente utilizzate laddove servono, cioè per le politiche attive del lavoro, per far sì che ci sia un incontro tra domanda e offerta di lavoro. Lavoro, questo sconosciuto. In questi giorni si è parlato tantissimo di Costituzione. A volte ci sorge il dubbio che non tutti la leggano fino in fondo. Porto qualche esempio. L'articolo 2,

Sì, però, chi è inabile al lavoro. Torna sempre quel concetto. Laddove non c'è la possibilità, si aiuta; laddove c'è la possibilità, ciascuno ha il dovere di svolgere il proprio compito. In sintesi, i diritti ci sono e vengono garantiti per tutti se ciascuno fa il proprio dovere. In conclusione, rivolgo gli auguri di buon lavoro al ministro Giorgetti, a tutti i membri del Governo e a tutti noi, senatrici e senatori di maggioranza ed opposizione. Il periodo è difficile, certo. A maggior ragione, tutti dobbiamo fare il nostro dovere.

In effetti il quadro economico è complicato. C'è una crisi energetica che si è attenuata, ma continua a mordere; c'è un'inflazione che ha rallentato, ma rimane molto alta (il carrello della spesa a marzo era oltre il 12 per cento); ci sono i tassi di interesse che sono molto aumentati e questo impatta sul debito pubblico, ma anche sui bilanci delle imprese e delle famiglie. I conti pubblici vanno meno bene di quanto dicono in apparenza i numeri del DEF e l'economia rallenta. Signor Presidente, ho visto tanta enfasi da parte della maggioranza per una crescita che quest'anno non sarà dello 0,6 per entusiasmo per uno zero virgola, come se fossimo in un *boom* economico. Ricordo che nel 2022 il PIL è aumentato del 3,7 per cento e nel 2021 del 7 L'anno prossimo peraltro - altro elemento di cui bisogna tenere conto - torneranno le regole di bilancio europee, di cui parleremo più diffusamente. La proposta della Commissione è un passo in avanti; lo ha detto correttamente anche il Ministro. Il commissario Gentiloni ha fatto un lavoro importante *(Applausi)* e credo che il Paese debba sostenere l'azione del commissario che esprimiamo, ma naturalmente quelle regole comporteranno dei vincoli che non avevamo nella fase di disattivazione delle clausole europee. Qual è il punto, però, signor Presidente? È che questo DEF non è prudente;

ha evocato la legge di bilancio per il 2024. Signor Presidente, servirebbero per la prossima legge di bilancio di legislatura da 25 a 30 miliardi di euro per fare il minimo sindacale: 10 miliardi per prorogare il cuneo fiscale; 5 miliardi per lasciare il finanziamento della sanità almeno al livello di quest'anno; i soldi per la scuola, i soldi per la riforma fiscale e i soldi che non ci sono per il contratto del pubblico impiego. Da 25 a 30 miliardi: questo DEF ne mette a disposizione quattro e per il solo 2024. C'è tanta propaganda nelle parole del Governo. Il punto è che non c'è una strategia per affrontare di petto i nodi della crescita e dello sviluppo, di quella mancata crescita e mancato sviluppo che invece, se affrontati, permetterebbero di allargare i margini di manovra della politica economica. Pensiamo al tema della doppia transizione, quella ecologica e quella digitale. Non è un tema per futurologi, perché le conseguenze del riscaldamento globale le stiamo pagando adesso: basta pensare ai danni della siccità, degli eventi climatici estremi. estremi. Dobbiamo prepararci per tempo alle conseguenze dell'automazione e dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sul nostro modo di studiare e di vivere. La politica, anche quella che scrive il DEF, dovrebbe comprendere la portata di queste trasformazioni e dovrebbe impostare per tempo le risposte. Qual è la risposta del Governo alla transizione ecologica? Avete fatto muro contro tutto quello che veniva avanti in Europa: muro contro il superamento dei motori a benzina e diesel dal 2035; muro contro la direttiva sull'efficientamento energetico degli edifici; muro contro tutte le scelte concrete che vanno verso la decarbonizzazione. Presidente, è che dietro questi muri c'è il vuoto totale; non c'è una politica industriale per accompagnare le nostre aziende e i nostri lavoratori di fronte alla transizione. *(Applausi)*. Lo abbiamo visto sull'*automotive*, su cui avete portato acqua alla Germania; avete fatto la battaglia sui biocarburanti e quegli altri hanno portato a casa i carburanti sintetici; voi, invece, non avete portato a casa l'unica cosa che serviva, non tempo, ma soldi spazi per una politica industriale che accompagnasse le imprese e i lavoratori italiani. Manca anche una politica industriale per cogliere le opportunità della doppia transizione, di nuovi posti di lavoro e nuove imprese. Avremmo bisogno di un nuovo piano Industria 4.0. Avremmo bisogno di mettere a terra i progetti del PNRR. Avremmo bisogno di una politica per lo sviluppo che non c'è in questo Documento di economia e finanza. Non c'è quella politica, ma abbiamo un Governo che continua a illudersi e a illudere gli italiani che si possa andare avanti con una competizione al ribasso. C'è il sommerso, e va bene, tolleriamolo; ci sono l'evasione fiscale, il lavoro sottopagato, la precarietà, di investire il meno possibile in ricerca e sviluppo. Questo modello di sviluppo che voi state portando avanti non ci porta da nessuna parte e in sei mesi sul PNRR, che era ed è l'occasione per cambiare questo stato di cose, voi avete perso tempo in chiacchiere. *(Applausi)*. Avete continuato ad annunciare una revisione del Piano di cui non c'è traccia a Roma e a Bruxelles e ieri lo abbiamo visto nelle parole del ministro Fitto. La verità è che voi non siete pronti, non avete chiaro quali progetti tenere e quali progetti spostare, quali procedure migliorare e come uscire dal pantano in cui vi siete messi. Il secondo nodo, Presidente, sono le disuguaglianze, che minano la coesione, ma rallentano anche la crescita. Nel 2022-2023 abbiamo avuto una fiammata inflazionistica che ha fatto crollare il potere d'acquisto dei redditi: cento di aumento delle retribuzioni, 8,7 per cento dell'inflazione, 12,1 per cento di inflazione per il 20 per cento più povero delle famiglie. È un carovita che allarga le disuguaglianze. Qual è la vostra risposta? 3,4 miliardi sul cuneo fiscale: una risposta che va nella direzione giusta, ci mancherebbe, ma con due limiti. Il primo limite è che sono pochi soldi: 15 euro al mese. Il secondo è che questo taglio termina a fine 2023 e non c'è un euro, non solo per prorogare il taglio del DEF, ma nemmeno per prorogare quello della legge di bilancio. però un problema ancora più serio: c'è una serie di decisioni che il Governo sta assumendo che va nella direzione sbagliata. Pensiamo alla riforma fiscale, che riduce la progressività e l'equità del sistema; pensiamo al no al salario minimo, al decreto lavoro che allarga il ricorso ai contratti precari, che smantella il reddito di cittadinanza, sostituendolo con strumenti che avranno il 30 per cento di risorse in meno. Pensiamo ancora a quello che il DEF non dice e ai soldi che non stanzia sulla sanità, che rischia il collasso con numerose Regioni che vanno verso il commissariamento. Ciò vuol dire taglio dei servizi e aumento della pressione fiscale per milioni di italiani.

a tutti l'educazione di lasciarci ascoltare?

riunificando strumenti che prima escludevano milioni di incapienti e di lavoratori autonomi e noi abbiamo messo 6 miliardi di euro in più rispetto a quello che c'era prima. Il Governo Conte II e il Governo Draghi hanno destinato agli asili nido e ai servizi per l'infanzia 4,6 miliardi del PNRR. Adesso il ministro Giorgetti è venuto in Commissione preannunciando un'azione *shock* di riduzione delle tasse sulle famiglie con figli,

non quelle che aiutano a fare la propaganda. Volete stanziare più risorse per invertire la curva demografica? Benissimo, ma allora raddoppiate l'assegno unico *(Applausi)*, che va anche agli incapienti e a tutte le famiglie italiane. Volete aiutare le famiglie a fare i figli? Mettete a terra i progetti degli asili nido del PNRR. *(Applausi)*. Anziché alzare bandiera bianca, realizzate quei progetti e usate i poteri sostitutivi se i Comuni non ce la fanno, anziché arrendersi. Volete aiutare le famiglie? Mettete a terra i progetti dei servizi per gli anziani, ampliate i congedi parentali, fate le cose che servono per aiutare le italiane e gli italiani a fare più figli. Se volete dare una mano al Paese, fatela finita con uno scontro ideologico sull'immigrazione, che non ci porta da nessuna parte *(Applausi)*, perché le aziende italiane che hanno bisogno di assumere non guardano il passaporto delle persone che assumono, ma guardano se sono capaci e hanno voglia di lavorare. Abbiamo tante aziende che non trovano lavoratori e non possono aspettare quando diventeranno utili al lavoro i nuovi nati, nell'immediato futuro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su tutti questi nodi economici e sociali state dando risposte sbagliate, sbagliate, ideologiche o nettamente insufficienti. Contrasteremo questa politica, perché è una politica sbagliata per il Paese. E la contrasteremo astenendoci sulla relazione al Parlamento e votando contro la risoluzione di maggioranza. Ma lo faremo a partire dalle nostre controproposte, che abbiamo costruito dialogando con le altre forze di opposizione e firmando una risoluzione insieme al MoVimento 5 Stelle e all'Alleanza Verdi e Sinistra,

di un lavoro che vogliamo proseguire e allargare a tutti, per costruire una diversa politica economica, ma soprattutto un futuro programma di Governo per il Paese.

posti di lavoro nel 2023; una riforma del *bonus* edilizio, che finalmente prenda in considerazione la sostenibilità e in particolar modo l'importanza del rapporto tra competenza e cassa.

+2,6 miliardi di euro nel 2025. Questa è l'attenzione nei confronti del Fondo sanitario nazionale, con una controtendenza importante rispetto ai tagli del passato, rispetto alle previsioni negative che avete fatto voi e rispetto allo smantellamento smantellamento della sanità del territorio, dei dipartimenti di prevenzione, della sanità delle aree interne. Questo è quello che ci avete lasciato. Mi dispiace non sia presente il presidente Monti. Credo non sia uno sgarbo istituzionale parlare in sua assenza, ma il suo atteggiamento nei nostri confronti, guardando da questa parte come un professore che si rivolge a neofiti della politica e dell'amministrazione, non mi è piaciuto, caro Presidente.

il presidente Monti non sa che chi parla, chi sta da questa parte, chi compone le file del centrodestra, chi compone le file di Fratelli d'Italia ha un passato glorioso, viene dalle piazze, sì, ma poi ha frequentato le aule dei Comuni, delle Province e delle Regioni. *(Applausi)*. Porta qui un'esperienza qualificata. Abbiamo studiato e mangiato polvere per diventare classe dirigente, non ci ha regalato nulla nessuno. È per questo che non ho preso di buon grado gli attestati di stima del del presidente Monti, che ci ha trattato quasi come fossimo dei discepoli, neofiti della politica appena entrati, con la sorpresa che ha denunciato nei nostri confronti. Abbiamo sfatato dei paradigmi, paradigmi, per cui lo Stato assistenziale è passato a essere uno Stato con un sistema che tutela i dipendenti e chi lavora. Tre miliardi nel 2023 vanno al cuneo fiscale, all'abbattimento delle aliquote Irpef, al fattore famiglia; miliardi e mezzo nel 2024 saranno linfa vitale per la riforma fiscale. Questo è quello che stiamo mettendo in campo. Sul Fondo sanitario nazionale vi ho già detto. Noi non adottiamo misure emergenziali, non adottiamo le misure *shock* alle quali voi siete abituati, perché sempre con Governi di piccola, misurata e misera prospettiva. Noi abbiamo una prospettiva di cinque anni. Abbiamo bisogno - e questo abbiamo scelto di fare di mettere in campo misure programmatiche, strutturali, che durino cinque anni, che diano respiro e certezze, che ci rendano credibili nei confronti della parte produttiva del Paese e dell'Europa, laddove oggi stiamo discutendo il Patto di stabilità, laddove poi saremo giudicati sul DEF, laddove poi saremo giudicati in base alle misure che produrranno la NADEF a settembre-ottobre di quest'anno. Guardando e ascoltando molti di voi - lo dico perché spesso mi piace evocare delle immagini prese in prestito dalla mitologia classica - ho pensato

esperto nella *techné*, nell'arte della costruzione, che aveva studiato, si era applicato e, forse proprio perché si era applicato, era prudente e misurato nelle scelte, nella misura in cui decide di costruire delle ali di cera e di piuma per il figlio Icaro, che voleva volare in alto e tornare ad Atene, uscendo dal labirinto; gli chiede di non volare troppo in alto e di non andare troppo vicino al sole, perché si sarebbero sciolte quelle ali, sarebbe caduto a terra e sarebbe morto. Ebbene, voi in questo volo siete stati per noi Icaro, che, nel tentativo di sognare troppo in alto con misure *shock* (superbonus e PNRR), siete andati al di là delle responsabilità e delle caratteristiche possibilità della nostra Nazione. *(Applausi)*. a fare il passo più lungo della gamba, a non avere contezza e consapevolezza dei nostri mezzi, dei nostri limiti e delle nostre possibilità. è arrivato il Governo Meloni, un Governo di centrodestra, a salvare la Nazione dal precipizio nel quale ci stavate portando. *(Applausi)*. Lo stiamo facendo con forza. Lo stiamo facendo con convinzione. Lo stiamo facendo guardando innanzitutto dentro noi stessi, nella consapevolezza dei nostri limiti e delle nostre misurate azioni. Noi siamo persone che, passo dopo passo,

con orgoglio, convinzione, riconoscenza nei confronti del ministro Giorgetti e gratitudine nei confronti del presidente Meloni e di tutto il Governo annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla risoluzione del Governo.

n. 243 del 2012. Avverto che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

ha deciso di non partecipare alle votazioni dei consigli di presidenza sulla giustizia amministrativa, sulla giustizia tributaria e sulla Corte dei conti. PRESIDENTE. Prego, senatore grave rottura, non solo delle prassi, ma anche di tutti i precedenti, come lei sa, e le do atto pubblicamente di aver provato a fare più volte una mediazione che sarebbe stata nell'esclusivo interesse delle istituzioni che rappresentiamo. Il Partito Democratico non parteciperà al voto perché non è mai successo fino alla giornata di oggi che la maggioranza decidesse anche per l'opposizione. Nei due precedenti che abbiamo alle spalle del 2013 e del 2018, i numeri che avevano portato poi alla definizione delle scelte dei consigli di presidenza erano stati rigorosamente rispettosi dei pesi dei Gruppi parlamentari; anzi, in un caso, nel 2013, addirittura la maggioranza di allora aveva dato più spazio alle opposizioni del tempo. In questo caso, signor Presidente, non solo la maggioranza ha deciso per l'opposizione,

Prendiamo atto della decisione della maggioranza di far diventare questa una vicenda che, di fatto, dà un profilo molto chiaro e, cioè, che non frega nulla - mi scusi, signor Presidente - alla maggioranza del quadro generale e del rispetto delle istituzioni.

mi corre l'obbligo di ricordare, avendo perfettamente compreso il suo intervento, che l'obbligo della parità di genere - obbligo, non opportunità è previsto per il CSM e non per tali organi. Capisco però il senso del suo intervento e la ringrazio per avermi dato atto degli sforzi degli sforzi che a qualcosa hanno portato qui al Senato. Capisco che voi vorreste un discorso complessivo che coinvolga Camera e Senato, ma io faccio il Presidente del Senato e voi siete senatori. Qui il rispetto dei precedenti c'è, perché

professor Alessio Lanzi I nomi sono pervenuti con regolare lettera sottoscritta ufficialmente dai Capigruppo, che rappresentano una larga maggioranza. Ricordo che in base alla citata disposizione di legge i due candidati saranno proclamati eletti se la lista posta in votazione otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea, cioè 104 voti. I senatori favorevoli alla lista proposta voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza. Dichiaro aperta

ciascun senatore riceverà una scheda di colore giallo, sulla quale indicherà un solo nominativo. Sarà proclamato eletto colui che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Per l'elezione dei due componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti, ciascun senatore riceverà una scheda di colore celeste, sulla quale indicherà sulla quale indicherà un solo nominativo. Sarà proclamato eletto colui che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Dinanzi al banco della Presidenza sono state predisposte due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti entrambe le schede, che dopo il voto depositeranno nell'apposita urna, all'uscita della cabina. La chiama sarà svolta in ordine alfabetico.

dei conti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, invito tre senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti. Subito dopo la

mi par di capire, dalla situazione, che sarebbe opportuno, intanto che si procede allo spoglio di questa prima votazione, che la seconda votazione venga rinviata

Apprezzate le circostanze e anche in ragione di quello che sto per dirvi, non procederemo adesso alla prevista votazione, che rinviamo a domani perché, non perché, non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta sulla risoluzione al DEF presentata alla Camera, a differenza di quanto avvenuto invece al Senato dove è stata raggiunta appieno la maggioranza prescritta, il Governo ha ritenuto opportuno, se non necessario - forse necessario, forse solo opportuno - riconvocarsi per

alla Relazione sullo scostamento, benché noi abbiamo regolarmente votato e approvato con i numeri prescritti, dovremo rivotare la nuova Relazione

poi si passerà alla votazione a maggioranza assoluta per l'eventuale approvazione; dopodiché la votazione che non abbiamo svolto ora, la faremo in coda, cioè non prima

Sarà una votazione con il sistema elettronico se nel frattempo avremo un accordo generale delle opposizioni o, comunque, si deciderà di presentare una lista

Mi pare di avervi detto tutto. Non ho altro da aggiungere se non augurarvi un veloce rientro a casa con ripartenza domani mattina